venga spiegato esattamente cosa è accaduto nella seconda parte della giornata, perché non si capiscono i meccanismi, la discussione e i motivi per cui si è operato il rinvio in Commissione. Io chiedo, sinceramente,

Fenu. Il Presidente, preso atto dell'orientamento espresso dai rappresentanti dei Gruppi, rinvia il predetto emendamento alla competente Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento.

senza tornare in Commissione e senza presentarne un altro. Il tema è proprio questo. Si è tentato, dal mio punto di vista,

Visto che da questo verbale non emerge il tentativo fatto dal relatore...

L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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

e io voglio capire cosa è successo. Ripeto, voglio capire dal relatore e dal rappresentante del Governo che cosa è successo. Forse i piaceri che dovevate fare, forse è arrivata una manina o una manona riguardo ad Autostrade.

Signor Presidente, io non voglio polemizzare e l'ho anche precisato, ma credo che il suo atteggiamento meriti le nostre attenzioni. Io chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di dare delle spiegazioni precise all'Assemblea e al Paese rispetto al loro atteggiamento: cosa è successo da ieri sera a stamattina? Vorremmo sapere dal Sottosegretario da chi è stato chiamato, persona che evidentemente non era soddisfatta completamente dall'emendamento presentato. Lo vorrei sapere, e non faccia lo spiritoso, dica delle cose serie. Lei ha fatto bloccare i lavori dell'Aula su un provvedimento così importante

sul decreto-legge fiscale sanno benissimo che l'emendamento girava nei banchi ormai da più di una settimana. È stato visto e rivisto, non era ancora stato presentato ma era ben conosciuto; quindi, non era assolutamente una novità. L'urgenza - su richiesta del Ministero - ha fatto sì che il relatore lo presentasse durante la giornata di ieri per una valutazione, sapendo benissimo che i lavori sarebbero proseguiti anche nella giornata odierna.

ovviamente nel rispetto del ruolo dell'opposizione, l'emendamento verrà presentato dal Governo in sede di legge di bilancio e quindi avrete tutto il tempo di valutarlo.

Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione l'intervento e le osservazioni svolte dal Capogruppo del Partito Democratico,

non è assolutamente possibile l'atteggiamento che avviene in questa Assemblea di mancanza di rispetto non soltanto nei confronti delle istituzioni ma degli italiani. Un emendamento come quello

ritengo, però, che sia difficile mettere in discussione un diritto costituzionalmente garantito e regolamentare della maggioranza di presentare emendamenti in Assemblea attraverso il relatore e ugualmente, nel momento in cui

emendativa è una necessità che abbiamo per intervenire su alcune infrastrutture di questo Paese che sono state abbandonate da un'incuria infrastrutturale che è sotto gli occhi di tutti. *(Applausi

Signor Presidente, anche io mi riallaccio agli interventi precedenti. È vero che è diritto del Governo e della maggioranza presentare e ritirare emendamenti si ha anche diritto a essere poco seri, ma sarebbe meglio non esserlo. Questo emendamento era già stato presentato in Commissione tardivamente;

disegno di legge di bilancio; corre altresì voce che questo intero testo, il decreto fiscale, con i suoi numerosi articoli e i numerosissimi provvedimenti che si sono aggiunti in corso d'opera, mettendo in grave

tutto nell'ambito del diritto (non ne sono neanche così sicuro), ma di certo non è nell'ambito della serietà. Il punto non è tanto il rispetto per questo o per quello, ma che ci sono delle procedure parlamentari per cui le decisioni vengono prese con trasparenza, in modo che chi ci osserva o chi viene a indagare sui lavori parlamentari una volta conclusi possa capire come e chi ha votato il provvedimento. decreti-legge che confluiscono in un altro provvedimento, emendamenti presentati, ritirati, ripresentati e nuovamente ritirati, la trasparenza che tanti invocavano mi sembra che venga gravemente pregiudicata e sicuramente è pregiudicata la serietà.

non vorrei che il fatto di aver aperto l'Assemblea con un po' di vivacità ci faccia perdere di vista le parole esatte del rappresentante del Governo, il quale ha

nella legge di bilancio, data la sua portata, mentre ieri sera si è chiesto di subemendarlo in mezz'ora, presentandolo dopo il termine che era stato stabilito per la chiusura dei lavori. Mi fa piacere se l'atteggiamento del Governo e della maggioranza è di ritorno alla serietà; lasciamo però agli atti che, se non fosse stato per una nostra battaglia, sarebbe stata stravolta una procedura che va nel rispetto dei lavori dell'Assemblea, quella di concedere tempi adeguati per subemendare

Presidente, intervengo solo per soddisfare il bisogno di approfondimento sull'accaduto evidenziato dalle minoranze. Vorrei solo portare due elementi fattuali che forse possono rassicurare circa eventuali intenzionalità politiche recondite che sono state evocate.

in Commissione - il capogruppo D'Alfonso me ne potrà dare atto - tutte le volte che un emendamento viene presentato si danno termini congrui per la presentazione di subemendamenti, ma in Commissione non era stato presentato alcun subemendamento a questo emendamento. Quindi quest'ultimo non era stato ritirato certo

Dal punto di vista procedurale, la Commissione ha fatto quello che poteva e doveva fare. Attualmente il tema mi sembra riguardi riflessione sulle coperture per un intervento la cui logica credo sia ampiamente condivisa e la cui necessità ci è stata sottolineata in Commissione anche dall'opposizione, perché il tema delle infrastrutture credo che comunque dovrebbe unirci e non dividerci. Tutto qui. Vi ho dato due elementi tecnici: dell'articolo 81 della Costituzione, ed è il motivo per cui l'emendamento è stato ritirato; quando è stato presentato in Commissione, sono stati dati tempi congrui e non sono state presentate proposte subemendative. Comunque grazie per questa opportunità di chiarimento.

Presidente, credo che la sorte di questo emendamento somigli a quella di Gian Burrasca, che compare e scompare. di un emendamento che fronteggia una questione reale, però richiede un metodo, che definisco di coltivazione, che deve tenere da conto

e consente la possibilità di continuare a mettere in servizio macchine per il gioco elettronico assolutamente sicure

che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni rilasciate dal MEF, sono necessariamente collegati

per gli apparecchi di cui al citato articolo 110 non possono essere più rilasciati dopo il 31 dicembre 2018. Ecco il motivo della proroga che

per la nuova generazione degli apparecchi per il gioco. La proroga è necessaria per garantire non solo entrate erariali, che altrimenti diminuirebbero visto il numero di macchine davvero sicure che verrebbe meno,

voglio intervenire in ragione di un importante emendamento che abbiamo presentato ed illustrato con attenzione, coinvolgimento culturale e - vorrei dire - anche storico in Commissione.

consistenza dal punto di vista dell'imponibile reddituale. La rendita INAIL fa, infatti, seguito a un pezzo di salute e di vita della persona che si è perso,

Giuridicamente, negli anni Sessanta e Settanta, dei giganti del diritto del lavoro hanno fatto in modo che le rendite INAIL venissero tolte dalla base imponibile; c'è stata poi leggerezza e superficialità e si è prodotta la consistenza in sede normativa sul piano della base reddituale delle rendite INAIL. Dobbiamo a tutti i costi recuperare il principio del diritto del lavoro di coloro i quali, per anni, hanno dovuto anche espatriare alla ricerca del lavoro. Pensate alle famiglie di coloro i quali hanno perso la salute a Marcinelle, ma

Non è assolutamente giustificabile e considerabile che il diritto positivo delle persone si genufletta nei confronti di una siffatta stravaganza intervenuta in sede di legiferazione, quando si è determinato che la rendita INAIL facesse

evitiamo però su questi argomenti il tentativo di scavalcare il momento nel quale si è creata concentrazione. Facciamo in modo che su questo si determini rimedio.

hanno riconosciuto ed evidenziato la necessità di rimediare. Ho difficoltà a parlarne poiché molti del mio paese di origine hanno dovuto purtroppo convivere

dal 1° gennaio 2019 - quindi, tra pochi giorni - dovranno pagare tutte quelle sospese, nonché quelle successive. Ciò significa - è giusto ribadirlo ancora una volta, soprattutto a chi ha fatto promesse elettorali, di cui fra un attimo

Sono oltre 200 i Comuni italiani che non hanno nemmeno un negozio e oltre 500 quelli che hanno un solo esercizio commerciale. In generale, la desertificazione commerciale è in crescita e - cosa molto più grave - ciò comporta poi la desertificazione residenziale nei piccoli Comuni con meno di 1.000 abitanti e in quelli di montagna. Il nostro emendamento nasce proprio con la finalità di salvaguardare i negozi sotto casa, il commercio di prossimità nei piccoli Comuni e nei centri delle aree montane. In quelle zone un negozio diventa, di fatto, una necessità sociale indispensabile, un vero e proprio ancoraggio ancoraggio della comunità, un luogo di aggregazione prima ancora che di acquisto, oltre che punto essenziale di servizio per i turisti. Tra l'altro, in diverse zone montane sono proprio i giovani che oggi, in controtendenza, non volendo abbandonare la propria terra di origine, scelgono di aprire imprese e attività commerciali, avviare *start-up* e *new-co* soprattutto nei settori del turismo, dell'agricoltura e della *green economy*, credendo fortemente nel rilancio dei territori montani e di quelli un po' più spopolati. Quindi, siamo di fronte a un ritorno alla tradizione, con nuovi sistemi che rappresentano la vera innovazione. occorre individuare delle misure fiscali vantaggiose, differenziate e peculiari per gli esercizi commerciali e le imprese presenti nelle aree montane e interne del Paese, così da compensare

IMU e TASI, a carico dei locatori o conduttori. Si tratta di comunicazioni che in realtà sono già note all'Agenzia delle entrate e, quindi, di una comunicazione annuale che potrebbe essere tranquillamente eliminata. Successivamente chiediamo un'armonizzazione dal punto di vista normativo, e cioè una definizione più stringente di ciò che è abitazione di lusso. A questo riguardo riteniamo che la normativa di riferimento dovrebbe essere il decreto ministeriale 2 agosto del 1969 e ciò perché, soprattutto per gli immobili di categoria A1, molte volte vengono indicate come di lusso abitazioni che non lo sono. Credo, quindi, quindi, che una piccola ricognizione di questi elementi, in Italia, ci consentirebbe di avere una normativa più attenta al riguardo. Poi si chiede la soppressione della comunicazione dell'anagrafe tributaria delle amministrazioni di condominio. Si tratta di obblighi che l'amministratore di condominio già svolge e sono già noti all'Agenzia delle entrate, per cui si tratta di un obbligo ridondante e inutile.

Berlusconi. Noi chiediamo che lo stesso regime sia consentito per gli immobili di proprietà condominiale. Ciò è possibile perché attraverso la ripartizione dei millesimi si dà la possibilità ai singoli proprietari di poter accedere a questa dichiarazione alternativa. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 20.0.200

di giornale sui terremotati abbandonati. Per brevità non cito tutti i problemi già risolti, dalle piccole difformità alle sanatorie pendenti a tutti gli interventi che sono stati fatti nei precedenti precedenti provvedimenti già approvati. Ricordo anche, per completezza, che nel testo iniziale non erano previste 60 rate e già le 60 rate sono una conquista introdotta da questo Governo. Da ultimo, è stato citato il terremoto del 2009, ma ci si è dimenticati

del Gruppo della Lega, ma che aveva anche l'adesione e il sostegno, ovviamente, del Gruppo MoVimento 5 Stelle, che auspicava la possibilità di valutare l'ulteriore aumento a 120 rate, compatibilmente con la sostenibilità del provvedimento. Non ci si può venire a dire, infatti, che bisogna seguire le indicazioni dell'Europa e stare stare attenti alle spese, e poi, dall'altra parte, proporre dei provvedimenti con dei costi notevoli, senza indicare come quei provvedimenti si intenda sostenerli sul piano economico. In conclusione, esprimo un voto contrario tecnico, ma di

potendo così avere un introito. È anche un modo per indurre i proprietari (stiamo parlando di grandi proprietà immobiliari) a mettere gli immobili sul mercato dell'affitto.

i proventi derivanti dall'incremento dell'aliquota ad interventi rivolti alla riqualificazione del patrimonio pubblico esistente.

l'articolo 20 è un articolo davvero pesante in questo decreto-legge, ragion per cui noi di Fratelli d'Italia, restando coerenti con la nostra proposizione costruttiva di un'opposizione che non vuole distruggere, che non vuole fare ostruzionismo ma che vuole proporre, nell'ottica di una crescita davvero felice (quella sì),

parlano delle zone logistiche semplificate per i porti del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, per Venezia e per Trieste; benefici fiscali, appunto, mirati a creare nuovi investimenti.

contribuenti che avrebbero portato imposte, da una parte, ricchezza e consumi, dall'altra, a tutto vantaggio del nostro PIL. Avevamo presentato emendamenti volti all'eliminazione di quella che era un'ingiusta gabella del populista Governo Monti, quella gabella che, dopo le tasse sugli *yacht*, aveva introdotto il superbollo sulle autovetture, sulle autovetture, che di fatto ha comportato la morte di un'intera area legata al commercio di autoveicoli, alla componentistica, ai meccanici, ai carrozzieri; che ha privato di un sogno i nostri giovani, i nostri cittadini che magari potevano utilizzare una macchina sportiva. Abbiamo, quindi, riproposto provvedimenti per i pensionati, per i cosiddetti pensionati al Sud modello Portogallo, quel modello che ha fatto recuperare al Portogallo un punto di PIL e che invece noi abbiamo beatamente ignorato.

quando ho avuto modo di spiegare la nostra disapprovazione sul fatto che siamo dovuti retrocedere, per pressioni probabilmente più alte di noi, su un punto importante quale la protezione, la tutela del credito nazionale, e nella fattispecie dell'unica banca rimasta italiana, com'è ancora oggi il credito cooperativo. Tutto questo, però, forse mi fa pensare che magari una nota positiva, almeno per la maggioranza, ci possa essere, ovvero una convergenza sui maggiori punti di questo decreto-legge *omnibus* tra la maggioranza grillo-leghista, da una parte, e il Partito Democratico, dall'altra. Amici miei, delle due l'una: se sulla fatturazione elettronica vi siete accodati ai Governo Gentiloni Silveri e al Governo Renzi, come sul tema dello Stato quale grande fratello fiscale, quella normativa che permette allo Stato di invadere, di conoscere le nostre risultanze finanziarie senza nemmeno ottenere l'assenso della procura della Repubblica, se su temi come il credito, appunto, vi siete accodati alla riforma Renzi-Padoan, se, cioè, su elementi pilastro, fondamentali, della precedente legislatura, in cui governava il Partito Democratico, voi della maggioranza grillo-leghista vi siete accodati, allora, vuol dire che presto farete un accordo e questo Parlamento avrà una maggioranza ben più ampia di quella che ha oggi. Questo è quello che tenevo a dire. Auspicherei un ravvedimento, me lo auguro in questa sede, quando voteremo gli emendamenti. Comunque, abbiamo ancora una prova d'appello, quindi mi rivolgo davvero di cuore agli amici e alleati della Lega: abbiamo una prova d'appello per il centrodestra, per il nostro popolo, nella legge di bilancio. Ricordiamocene; ricordiamoci dei nostri programmi elettorali, del nostro popolo, dei lavoratori autonomi, delle piccole imprese e votiamo coerentemente.

intervengo solo per chiarire un difetto di comunicazione con la Presidenza:

Grazie, L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Governo sulle decisioni in materia di bilancio». Ha facoltà di parlare il ministro dell'economia e delle finanze, professor Tria.

Signor Presidente, senatrici e senatori, svolgo a nome del Governo una comunicazione sul disegno di legge di bilancio attualmente in discussione alla Camera. anche riferire sull'intenso dialogo in atto con la Commissione europea sul quadro programmatico di bilancio che di tale legge è la base e sul quale la Commissione ha espresso una posizione critica. Un dialogo improntato a individuare una possibile soluzione condivisa nel pieno rispetto delle priorità di politica economica delineate dal Governo. Vorrei ricordare che il disegno di legge di bilancio in discussione declina la strategia del Governo di rilancio della crescita e dell'occupazione e di contrasto alla povertà attraverso una manovra fiscale moderatamente espansiva. Questa strategia muove dalla constatazione del basso tasso di crescita di cui ha sofferto l'Italia nell'ultimo decennio e, in particolare, come abbiamo più volte ricordato, dalla constatazione che esso è rimasto costantemente al di sotto di quello medio europeo di circa un punto percentuale. Ciò ha determinato il fatto che, dopo la crisi del 2008, oggi siamo ancora lontani dal livello del PIL di dieci anni fa, dal livello di disoccupazione di dieci anni fa e che, di conseguenza, è aumentata in modo insopportabile l'area della povertà e del disagio sociale, mentre, al contempo, non si è né raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito pubblico che pesa sull'Italia, né il pareggio di bilancio, cioè l'obiettivo di medio termine indicato dalle regole fiscali europee. In altri termini, non abbiamo ancora avuto una stabilizzazione né economica, né sociale, né della finanza pubblica. Oltre a ciò, voglio ricordare che si è materializzato, in misura sempre più netta nel corso del terzo trimestre, un rallentamento dell'economia europea e italiana che ci ha posto davanti alla necessità di un intervento teso a contrastare tale dinamica negativa da subito. In altri termini, all'esigenza di agire per un aumento strutturale del tasso di crescita si è aggiunta la necessità di attuare un'azione anticiclica di contrasto al rallentamento dell'economia. In questo quadro, la manovra posta in essere con il disegno di legge di bilancio in discussione alla Camera è stata disegnata per perseguire i due obiettivi fondamentali di natura economica sui quali il Governo si era impegnato fin dal suo insediamento: aumentare il tasso di crescita e ridurre, anche per questa via, il rapporto debito pubblico-PIL. I pilastri dichiarati della strategia del Governo diretta a conseguire questi obiettivi sono il rilancio degli investimenti pubblici, l'avvio delle riforme fiscali, il rafforzamento del contrasto alla povertà e delle politiche attive del lavoro e la riforma del sistema pensionistico allo scopo di eliminare i problemi di transizione creati dalla riforma Fornero. Ho più volte riferito in Parlamento i motivi per i quali tutte queste misure, anche quelle di spesa corrente più dedicate alla protezione sociale, devono concorrere a creare un contesto favorevole alla crescita, determinando le necessarie condizioni di stabilità e inclusione sociale. Per ciò che riguarda il quadro di finanza pubblica, ci siamo trovati, com'è noto, di fronte alla necessità Grazie,

secondo la risoluzione approvata da questo Parlamento in giugno, la clausola di salvaguardia relativa all'incremento dell'IVA pari a 12,5 miliardi indicata dal precedente Governo. La manovra programmatica si è quindi limitata ad aumentare per il 2019 il *deficit* tendenziale di circa quattro decimali al fine di finanziare misure che avessero, al contempo, effetti positivi sul potenziale di crescita di medio e lungo periodo del sistema economico del Paese e un effetto espansivo nel breve periodo. In questo quadro programmatico si è anche posto, in modo più deciso che nel passato, il rapporto tra debito e PIL su un sentiero di riduzione, seppur in misura ancora non soddisfacente. Siete a conoscenza che il bilancio programmatico che sostiene la legge di bilancio in discussione è stato tuttavia contestato dalla Commissione europea, con una prima richiesta di presentare un documento di programmazione del bilancio rivisto e che tenesse maggiormente in conto l'obiettivo di medio termine in merito alla riduzione del *deficit* e al percorso di riduzione del debito. Le obiezioni della Commissione si sono basate anche sulla contestazione della nostra previsione di crescita e, quindi, sull'evoluzione attesa del *deficit* e del debito. A questo proposito, tengo a ribadire ancora una volta che le previsioni di crescita programmatiche adottate dal Governo in settembre si basano su una stima metodologicamente corretta dell'impatto del maggior *deficit* programmato sulla crescita tendenziale, sulla crescita tendenziale, stimata in linea con quelle allora correnti. Le informazioni successive indicano un deterioramento più deciso delle prospettive di crescita, ma faccio osservare che le stime Istat, rilasciate successivamente, in novembre indicano per il 2019 un tasso di crescita che si discosta di soli due decimali (1,3 contro 1,5) da quello indicato in settembre dal Governo come conseguenza delle misure da adottare. Tuttavia, la risposta della Commissione europea al nuovo Documento di programmazione di bilancio, che è stato ripresentato in ottemperanza alle regole europee che sovrintendono al semestre europeo e al confronto comunitario, risposta ufficializzata il 21 novembre scorso, riafferma l'opinione iniziale di non conformità al percorso di aggiustamento strutturale verso l'obiettivo di medio termine raccomandato dalla Commissione, evidenziando una deviazione significativa da questo percorso. Questa opinione, se confermata dal Consiglio europeo dei ministri finanziari, apre la prospettiva di una procedura di infrazione per *deficit* eccessivo basata sul debito. Si tratta di una prospettiva che pone oggi il Governo e il Parlamento sovrano di fronte alla necessità di assumere decisioni di forte responsabilità nazionale, ma che, proprio per questo motivo, richiede anche una forte operazione di verità sulla quale costruire un ampio consenso. Quanto eccepito dalla Commissione europea - vorrei ricordarlo nella modifica sostanziale di quei fattori rilevanti analizzati dalla Commissione stessa il 23 maggio 2018, quando decise di non sanzionare il non raggiungimento da parte dell'Italia dell'obiettivo raccomandato di riduzione del debito. La decisione di non sanzionare l'Italia, infatti, fu presa in base al profilo di aggiustamento strutturale proposto dal precedente Governo per il triennio successivo 2019-2021, profilo chiaramente poco realizzabile, sorretto da clausole di salvaguardia fiscale di misura crescente nel tempo e ancora più non sostenibile in una fase di rallentamento dell'economia. Il Governo precedente si era quindi impegnato con la Commissione ad un percorso di aggiustamento del *deficit* e del debito italiano, prescindendo dal realismo del suo conseguimento. Il nostro bilancio programmatico non poteva quindi confermare quell'impegno e ha deviato per i motivi sopra esposti. La Commissione ha dunque rilevato che cadevano i presupposti della sua decisione di accettare come non deviante il livello del debito riscontrato per il 2017. Non si tratta qui di attribuire responsabilità a chi ci ha preceduto nella responsabilità di Governo, perché di fronte alla Commissione europea c'è lo Stato italiano, rappresentato dal Governo *pro tempore*, che quindi è tenuto a farsi carico di tutta la nostra storia. Ciò non toglie che dobbiamo chiederci per quale motivo ci troviamo oggi a doverci far carico di una situazione della finanza pubblica che ci pone in obiettiva difficoltà. Non possiamo dimenticare che l'Italia ha beneficiato della politica espansiva monetaria dal 2015, in particolare, del *quantitative easing*, che ha portato nel periodo 2014-2018 a un risparmio sulla spesa per interessi che può essere stimato in circa 35 miliardi di euro, risparmio che non si è riflesso in una discesa del debito né, se non solo molto parzialmente, in un contenimento del *deficit*. abbiamo invece avuto un aumento della spesa corrente, che ha assorbito tale beneficio, in gran parte per finanziare la stagione dei tanti *bonus*, che ha generato un onore che continua a pesare sul nostro bilancio.

anche nell'ultimo triennio, in cui la Commissione ha concesso la flessibilità di bilancio, al fine di aumentare gli investimenti pubblici. Soprattutto, è costantemente diminuita la capacità di programmazione e progettazione degli investimenti, che non ha consentito di sfruttare a pieno neppure le risorse che si sono rese disponibili nel tempo. Tutto questo ha portato l'Italia in una situazione contraddistinta dal consolidato ritardo di crescita rispetto alla media europea, che non ha consentito, neppure negli ultimi anni, di ridurre il peso del debito pubblico sulla nostra economia. Come già detto, non è nostra intenzione parlare di responsabilità del passato, nel momento in cui dialoghiamo con la Commissione europea, perché quella che ho ricordato è la nostra recente storia comune,

è affrontare problemi concreti, non certo organizzare un affronto all'Europa stessa o un'uscita dall'euro. Tuttavia, dobbiamo tener conto dei timori dei nostri *partner* europei del grado d'incertezza che pervade i mercati e il mercato finanziario in particolare, sia per l'incertezza sull'evoluzione dell'economia globale, sia perché preoccupano le divergenze con l'Europa. Soprattutto, dobbiamo tener conto dell'incerto contesto economico in cui ci muoviamo e dell'alto livello dello *spread*, che incide su tale contesto. Quando abbiamo un rallentamento dell'economia, si pone sempre un dilemma: da una parte si manifesta la necessità di rafforzare le misure di sostegno all'economia, anche se ciò implica un allargamento del bilancio; dall'altra, poiché la minore crescita si riflette negativamente sul bilancio pubblico, si pone il problema di una maggior prudenza di spesa. Si tratta di un dilemma che richiede un serio bilanciamento delle politiche adottate. Oggi, al dilemma richiamato, si sovrappone anche la necessità di non divergere da regole derivanti dai nostri impegni europei, nella misura in cui ciò rischia di produrre, di per sé, effetti negativi sulla crescita e sulla stessa politica espansiva che abbiamo deciso, facendo aumentare il costo del finanziamento del debito pubblico e, in prospettiva, del finanziamento dell'economia. È con questo spirito di ricerca dell'equilibrio che abbiamo costruito la nostra legge di bilancio e stiamo oggi dialogando in modo virtuoso con la Commissione per trovare miglioramenti condivisi, miglioramenti che il Parlamento può apportare nella sua sovranità.

Per parte nostra, abbiamo proposto di rafforzare l'obiettivo di riduzione del debito anche attraverso una mirata dismissione di attività pubbliche, ma il punto centrale è che dobbiamo dedicare ingenti risorse agli investimenti pubblici, investimenti nelle infrastrutture e nei territori, puntando ai settori strategici e alla messa in sicurezza. È necessario inoltre garantire un alto tasso di innovazione tecnologica incorporata in questi investimenti. Dobbiamo però anche tenere conto della preoccupazione della Commissione europea che richiama al rispetto delle regole, pur ribadendo una volontà di dialogo costruttivo con l'Italia. È infatti consolidando un clima di fiducia che potremo invertire le aspettative dei mercati, dei risparmiatori e dei consumatori, affinché gli effetti attesi dalla manovra del Governo si possano realizzare. Stiamo quindi attentamente valutando, man mano che il disegno delle principali misure viene tecnicamente definito e quindi sono più attentamente valutati i loro costi effettivi, se si possano trovare spazi finanziari per migliorare l'equilibrio tra la necessità di sostenere ancor più la crescita e la e la necessità di consolidare la sostenibilità dei conti pubblici. In questa direzione anche il dialogo con la Commissione europea ed i nostri *partner* europei può trovare spazi nuovi e condurre ai risultati che da entrambe le parti vengono auspicati. Signor Presidente, senatrici e senatori, questo è il quadro complessivo nel quale ci muoviamo; un quadro caratterizzato dalla volontà imprescindibile di agire in favore della crescita e dello sviluppo per garantire dignità e lavoro ai nostri concittadini, dalla necessità di ripristinare un contesto di fiducia rispetto alle nostre posizioni in Europa, dall'attenzione allo stato attuale della finanza pubblica e dal percorso di riduzione del debito. Questi profili caratterizzano sia la proposta del Governo, sia l'intenso negoziato in corso con la Commissione europea, sia l'interazione con il Parlamento, che rimane il luogo istituzionale dove i miglioramenti alla proposta del Governo possono essere realizzati e approvati. È mio più sincero auspicio che guardando ai fatti senza drammatizzazioni, ma con grande lucidità e responsabilità per il bene del Paese, potremo tutti insieme giungere a un esito che rappresenti la soluzione ottimale rispetto ai tre punti fondamentali che ho esposto. Lo faremo senza rinunciare alle nostre priorità. *(Applausi

di come sta procedendo e su quali basi si sta nei fatti articolando il dialogo con la Commissione europea.

Lei è venuto, Ministro, a ricordarci quali sono gli assi su cui avete confezionato la manovra di Governo. È una discussione che abbiamo già affrontato nell'ambito della Nota

europea. Da oltre due mesi, di fatto, la politica e l'economia dell'Italia ruotano intorno a due riforme: la parziale revisione della riforma Fornero e il cosiddetto reddito di cittadinanza.

di lotta alla povertà e di aiuto al reddito; ma per assicurarsi, Ministro, una possibilità reale di ripresa del Paese e di aumento del tasso di crescita è indispensabile una forte manovra di investimenti pubblici.

virata della manovra stessa per spostare almeno una parte del *deficit* sul piano degli investimenti. Gli investimenti certamente non possono essere casuali e hanno la necessità

voi avete mai forzato? Siete andati in Europa a dire che non ci state a queste regole? Avete posto una questione per cambiare le regole? Noi siamo contrari ci batteremo fino alla fine per rivedere il *fiscal compact*, ma quando si va in Europa, ancor prima di presentare la manovra in *deficit*, si deve avere il coraggio di dire che le regole, seppure non le forziamo, le vogliamo cambiare. La prima questione da porre era quella di

Oggi lei è venuto qui a spiegarci quanto è bella la vostra manovra, ma non ci ha voluto spiegare quali sono gli assi su cui state portando avanti il dialogo. Io sono molto franca:

ancor di più vale il fatto che quello 0,2 non deve andare in riduzione di per sé del *deficit*, ma dovrebbe essere utilizzato per un piano di investimenti. Come voi siete prigionieri

Quella manovra così com'è, proprio perché non presenta nulla di serio, concreto e nuovo sul piano degli investimenti e quindi di una politica che possa davvero far crescere il Paese,

Che cosa dovremo dire alla fine delle sue comunicazioni? Finalmente i toni sono stati gentili e si apprezza il dialogo, ma ancora una volta non si comprende quali sono gli assi fondamentali su cui si vuole procedere nel rapporto con la Commissione europea.

Signor Ministro, lei e il suo Governo state per entrare nei libri di testo di economia. Il problema è che state per diventare un caso di studio esemplare di una nuova fattispecie di politica economica: una politica economica espansiva con effetti recessivi, un vero capolavoro. Fate nuovi debiti, aumentate il PIL programmatico di 1, 2 punti rispetto al tendenziale peggiorate il *deficit* strutturale di quasi un punto percentuale, ma le stime dell'Unione europea parlano di numeri e stime ben maggiori, cui voi non state rispondendo (non lo ha fatto oggi neanche lei,

trovare i soldi. Risorse del bilancio pubblico saranno dirottate da impieghi produttivi alla spesa sugli interessi. La Banca d'Italia ha parlato di un costo dello *spread*, in termini di spesa degli interessi sul debito, pari a già 1,5 miliardi quest'anno, per arrivare - forse - a 5 miliardi nel 2019 e a 20 miliardi nel 2020. Insomma, state facendo una manovra espansiva, ma dagli effetti recessivi. E tutto questo per due motivi: il primo è il modo disordinato e autolesionistico con cui avete impostato il dialogo con l'Unione europea, isolando l'Italia rispetto a tutti gli altri Paesi; il secondo motivo è la visione, o - meglio - l'assenza di visione, che sta dietro alla vostra manovra di bilancio. Mi soffermo sul primo motivo. Per carità, con l'Unione europea si deve negoziare, anche in maniera dialettica, dicendo le cose che non vanno, è stato fatto dai Governi a guida del Partito Democratico, negoziando flessibilità di bilancio in cambio di riforme strutturali e investimenti per dare ossigeno a famiglie e imprese nel breve periodo e rilanciare la crescita potenziale nel lungo.

aiutando chi vuole scommettere contro l'Italia e, magari, chi tra un po' si vorrà prendere a saldi pezzetti di tessuto produttivo o bancario. Siete passati da toni bellicosi e proclami di guerra, con tanto di scarpe esibite sui tavoli e offese personali a chi rappresenta noi cittadini europei,

il vero problema non è l'Unione europea ma la vostra manovra. Il problema non sono gli zero virgola e i numeretti della legge di bilancio, bensì gli zero, le priorità sbagliate e le soluzioni che non ci sono: zero crescita, zero lavoro di qualità, zero sostegno alle famiglie con figli, zero sostegno alla non autosufficienza, zero investimenti (investimenti veri, non trucchi contabili).

come se la politica non si debba preoccupare di cosa succede tra dieci anni, del futuro del nostro Paese. Il futuro è la nostra vita, è il nostro benessere, è il Paese che lasceremo ai nostri figli (e ve lo dice qualcuno che, purtroppo, non ha figli). Il futuro è il motivo per cui si dovrebbe fare politica. Il futuro non è una discarica dove nascondere le scorie radioattive delle vostra incapacità di governo e delle vostre promesse irrealizzabili. Per la legge di bilancio individuate due priorità: il fantomatico reddito di cittadinanza e la pensione anticipata per tutti. Concludo dicendo che non individuate misure concrete neanche su queste due priorità. Fate dei fondi e tanti proclami sui giornali o su Facebook ma non ci sono le misure concrete. Create incertezza, create aspettative. Le risorse che sono in quei fondi non basteranno per fare tutto quello che state promettendo. Il problema non sono i numeretti di questa legge di bilancio. Il problema sono i vostri giochetti che mettono a repentaglio il benessere futuro delle italiane e degli italiani. Grazie, Signor Presidente, signor Ministro, è oggettivamente imbarazzante la scena cui abbiamo assistito con il suo intervento mentre i tanti mister Hyde del suo Governo vanno nelle piazze a propagandare un atteggiamento molto muscolare nei confronti dell'Europa, uno sprezzo sovrano e dignitoso di ogni attacco ricevuto dalle istituzioni e dai mercati, e rassicurano la popolazione sul fatto che tra breve pioverà denaro nelle tasche di tutti gli italiani, a cominciare giustamente e solennemente dai più poveri, poi arriva qui il dottor Jekyll che ci dice che vi siete accorti che forse qualche allarme che era stato lanciato anche dalle opposizioni responsabili e patriottiche come Fratelli d'Italia era vero. Non siamo cioè nel paese di Bengodi, abbiamo un fardello pesante (tornerò anche su questo), fase di recessione economica che sta colpendo l'Europa e il mondo, e l'Italia in questi decenni ha purtroppo sempre dimostrato che in tempi di recessione il suo PIL

nella Nota di aggiornamento al DEF avete avuto la presunzione di dire che, in previsione di una recessione in arrivo, l'Italia avrebbe non soltanto

accademica che se fosse riuscita sarebbe valsa il Premio Nobel per l'economia da qui ai prossimi dieci anni. La realtà, prima o poi, ci costringe a fare i conti. È che è in arrivo una recessione economica che inevitabilmente avrà un impatto sull'Italia, al di là della bontà del Governo e delle sue manovre, perché L'Italia sarà, sì, una grande economia ma è sempre troppo piccola di fronte all'economia globale per non dover subire le influenze di una recessione economica che coinvolge tutto il mondo e soprattutto il mondo occidentale e l'Europa di cui facciamo parte. È chiaro quindi che quando arriva una tempesta inevitabilmente noi ne subiamo Grazie,

non serve a niente - ed anzi è addirittura dannoso e controproducente - mettersi a fare la bega interna e scaricare la responsabilità sulla parte politica che ha governato ha governato prima di chi in quel momento rappresenta l'Italia, perché quando si è all'estero si rappresenta il Paese, bisogna saperlo fare e quindi è giusto assumersi la responsabilità di tutta la storia del proprio Paese, della propria Nazione. però siamo in Italia, siamo nel Senato della Repubblica e qui ci possiamo non soltanto permettere di raccontare, ma anzi è doveroso registrare quello che è accaduto e cioè che negli anni del *quantitative easing*, cioè dei soldi facili garantiti dalla Banca centrale, che avrebbero dovuto aiutare l'Italia a fare buona scorta e ridurre il *deficit*, abbiamo avuto invece Governi a guida del Partito Democratico che hanno sciupato quelle condizioni economiche. Lo hanno fatto facendo, peraltro, uno scambio, che noi criminale, tra accettare l'immigrazione incontrollata e avere quindi la possibilità riconosciuta dall'Europa di una maggiore possibilità di spesa, che oltretutto hanno sciupato ulteriormente non utilizzando i soldi e la flessibilità in più garantita dall'Europa in cambio della volontaria adesione all'invasione del nostro territorio e alla creazione di una bomba sociale, demografica e culturale dell'Italia che non sappiamo come affrontare. Poi c'è qualcuno che oggi si deve fare carico delle promesse di rimpatriare 600.000 immigrati clandestini che non possono essere

ha una gravissima responsabilità. Badi bene, però, signor Ministro, che sostituire i piccoli *bonus* da 80 euro - per raccontarne solo uno - con il mega-*bonus* del reddito di cittadinanza non è una politica tanto diversa

in maniera più o meno dignitosa, in piedi piuttosto che in ginocchio, per ottenere un altro margine di flessibilità, lo si brucerà, invece che per diminuire il debito e raddrizzare la bilancia dei pagamenti (mediante politiche di crescita e di sviluppo economico attraverso il taglio delle tasse, la semplificazione burocratica, gli incentivi veri alla crescita economica e a chi dà lavoro), per fare questi *bonus.* Poi la prossima volta ci ritroveremo un Governo che avrà fatto delle promesse e avrà inserito clausole di salvaguardia pesantissime, che prevedono per i prossimi anni tassazioni esorbitanti e intollerabili, e ciò naturalmente pregiudicherà il futuro dell'Italia. Signor Ministro, noi avevamo detto esattamente queste parole quando abbiamo dovuto discutere della politica economica all'inizio della manovra di bilancio, in occasione dell'esame della Nota di aggiornamento al DEF e poi già alla Camera

per fare investimenti infrastrutturali seri che rilancino l'economia e non per buttarli nel reddito di cittadinanza e in altre spese correnti

e cercate di capire quello che sta avvenendo e qual è il rischio cui state esponendo il Paese». Signor Presidente, Ministro, colleghi senatrici e senatori, siamo al tedioso e ripetitivo teatrino: il valzer di numeri di questa manovra e delle sue misure, infatti, non sembra arrestarsi Tra un vertice e l'altro, a Palazzo Chigi, sulla manovra riprendono le girandole dei comunicati, delle interviste nei *talk-show*, delle smentite, dei *tweet*, delle dirette Instagram, dove si dice che i saldi non cambiano, che i decimali non si limano o ancora che non ci si attacca ai decimali ma che le misure non si ritardano; che le iniziative non si annacquano, che continuerete a tirare dritto. A starvi dietro si fa un'enorme fatica, e ci sta: il mestiere dell'opposizione è cosa impegnativa è seria, si sa, ma qui di poco serio - mi spiace dirlo, signor Ministro, proprio a lei, che invece spesso appare quasi isolato nel dimostrare senso delle istituzioni e rispetto nei confronti degli impegni assunti - c'è il vostro insieme, che risponde al nome di «compagine di Governo». Il famoso gioco del poliziotto buono e del poliziotto cattivo - a proposito, leggevo giusto ieri che la figlia di Salvini pensa che il padre faccia il poliziotto, guarda caso! - o ancora meglio la tecnica del bastone e della carota sono talmente abusati dai principali azionisti dell'attuale Esecutivo che il precipitato reale di questa vostra dialettica si polarizza in una secca perdita di credibilità del nostro Paese. Volerete nei sondaggi, forse, o forse immaginate di riuscirci raccontando bugie, ma gli osservatori internazionali, i *partner* europei, gli investitori hanno ormai espresso a più riprese un giudizio critico. Avete deciso, infatti, di mettere in piedi un teatro dell'assurdo a ciclo continuo, dove va in scena - da mesi ormai - un'opera che sta demolendo quei segnali di ripresa che si susseguivano da ben quattordici trimestri - ripeto, quattordici - senza soluzione di continuità. Ebbene, avete spezzato il giro e lo state facendo pagare con i risparmi degli italiani. È un prezzo, questo, doppiamente insopportabile perché mette in fibrillazione il presente per via della impennata che ha segnato lo *spread* e si traduce in un'ipoteca pesante che verrà riscossa nel prossimo futuro. Per questo oggi, signor Ministro, il suo intervento in Aula ci ha deluso, perché speravamo assumesse una diversa rilevanza, un approccio diverso. È stata una relazione, la sua, oggettivamente imbarazzante. Con la risoluzione che il PD ha presentato, volevamo aiutarvi a costruire un argine, un saggio perimetro di contenimento per la salvaguardia dei risparmi degli italiani, e, tramite questo, mettere al riparo anche l'accesso al credito, con buona pace dunque di quelle nuove teorie economiche lanciate dalla viceministro Castelli per la quale lo *spread* non influisce sui tassi dei mutui. come se non fosse già abbastanza, la questione *spread* è, purtroppo, solo una parte di quel Moloch che avete messo insieme con la vostra legge di bilancio. Avete disegnato e immaginato la manovra senza la minima considerazione del contesto macroeconomico in cui va ad insistere. Non avete preso in minima considerazione i segnali di indebolimento dell'economia, con una minore crescita stimata da ISTAT sia nel 2018 che nel 2019 e nel 2020. Lei li ha citati anche oggi qui, ma non ne avete voluto tener conto. Come fanatici totalitaristi, continuate a pensare che il consenso del 4 marzo sia più forte della realtà e che quindi volere è potere, punto e basta. Il tutto, poi, come sempre, condito da una retorica semplicistica e *naïf* che solo oggi, o meglio da un paio di giorni, vediamo tenuemente venire sconfessata, *in primis* proprio dall'avvocato del popolo, il professor Conte, e pur tuttavia non convince nessuno. La sensazione è che l'obiettivo di Salvini e Di Maio sia solo quello di arrivare alle elezioni europee senza sanzioni, puntando ad allungare i tempi della procedura UE di infrazione, che di fatto è già stata avviata. Al tavolo dell'Esecutivo, riuniti a più riprese per discutere sulla manovra, la maggioranza resta sempre più divisa:

visto che USA e Germania sono nel nono anno consecutivo di espansione e visti i rischi protezionistici - l'Italia non avrebbe più spazio fiscale per combattere la recessione ed evitare gravi conseguenze su redditi, occupazione e povertà. la questione sul tappeto non è da poco. Il quadro di finanza pubblica che si delinea in base alle scelte individuate dal Governo non solo è imprudente, in linea di principio e in prassi neanche sostenibile, perché le iniziative che avete scelto di finanziare in *deficit* non sono neanche inserite nella norma. Una su tutte: il reddito di cittadinanza. Affermate che con il reddito di cittadinanza ripartiranno i consumi, ma il modo con cui lo state costruendo è - a voler essere buoni una scommessa su una promessa insostenibile: attribuite effetti espansivi ad un'iniziativa che di fatto continuerà a non esistere anche quando la manovra sarà legge. Altro che finanza creativa, signor Ministro, qui siamo ben oltre! Fermatevi, forse siamo ancora in tempo.

a parlare di legge di bilancio e a cercare di spiegare qualcosa che tutti noi avevamo e abbiamo letto sui giornali o abbiamo ascoltato dalla radio o dalla televisione. Le debbo dire che probabilmente ho capito che prima di tutto vi è una sua personale soddisfazione

la sua soddisfazione per avere avuto probabilmente ragione di nutrire quella preoccupazione che, nei vari convegni e nei momenti

fa parte. Signor Ministro, cari colleghi, emerge un dato dopo alcune settimane, dopo aver bruciato circa 70 miliardi di euro di capitalizzazioni, dopo che il sistema europeo - non soltanto la Commissione ma anche quanti erano reputati nostri amici all'interno dell'Unione europea - ci ha puntato il dito esser stati richiamati da tutti gli organismi internazionali che guardano con attenzione al sistema economico europeo,

le due componenti di questo Governo avevano sostenuto, da una parte, il reddito di cittadinanza come la soluzione ai vari problemi di povertà di questo Paese e che, dall'altra parte, la Lega aveva sostenuto che con quota 100 avremmo risolto i problemi dei pensionati italiani che giustamente dopo l'età di sessantadue anni, o i trentotto/quaranta anni di lavoro dovevano andare legittimamente in pensione. Ebbene, dopo tutto questo, dopo la legittima difesa del rapporto con il proprio elettorato, oggi lei ci dice che questa è una manovra moderatamente espansiva, che la nostra crescita è un punto e mezzo sotto la media europea che probabilmente il *deficit* programmato dovrà essere ridotto, altrimenti l'Unione europea ci continuerà ad additare e a mettere sotto

che il suo punto di vista, *ante* approvazione della Nota di aggiornamento al DEF, era corretto, e che quello che le dicevano i suoi danti causa era sbagliato. Bene, il tema è proprio questo, e io lo dico agli amici del MoVimento 5 Stelle, lo dico agli amici della Lega: voi oggi prendete atto di una situazione (ed è un problema per (ed è un problema per gli italiani e non soltanto per voi): quella di non poter portare a casa quegli impegni che vi eravate presi con il cosiddetto contratto di Governo. Questo è il dato. Ma chi ci rimette non siete soltanto voi che - a questo punto emerge effettivamente e plasticamente - non siete in grado di portare a casa gli impegni che avete assunto, ma sono le famiglie e le imprese. Stiamo discutendo in quest'Aula da ieri e in Commissione da settimane del decreto-legge fiscale dove ci sono nuove tassazioni per le imprese, dove sono state cancellate o quasi le detrazioni fiscali e dove non ci sono incentivi per lo sviluppo: il problema è qui. il problema è qui. Intestardirsi per andare nella direzione di portare a casa due manovre come quelle che lei ha ricordato oggi, il reddito di cittadinanza e la quota 100, vuol dire impoverire questo Paese. questo Paese. Noi arriveremo ad avere un quasi reddito di cittadinanza, arriveremo ad avere una quasi quota 100, e stiamo arrivando ad avere una quasi legge di bilancio. Guardate che impuntarsi e intestardirsi in questa direzione vuol dire soltanto andare ad impoverire questa nostra Nazione. Noi ci eravamo presi un impegno, e lo dico agli amici che facevano parte della nostra maggioranza eletta dagli elettori il 4 marzo con 12.150.000 voti. Noi avevamo detto che avremmo abbattuto le tasse con una *flat tax* con aliquota unica; avevamo detto che avremmo previsto un'esenzione per le assunzioni fino a trentacinque anni di età per sei anni; avevamo detto che avremmo dato una soluzione vera alla povertà.

Lei doveva essere più esplicito, come regalo di compleanno. Lei doveva venir qua e dire: avevo ragione io, il Governo ha sbagliato; stiamo tentando di rientrare in un'impostazione che avevo dato; probabilmente non mi hanno capito e il futuro che abbiamo di fronte è buio, nero e pieno di buche. Quindi invito tutti gli amici della maggioranza a rivedere le proprie posizioni. Guardate che fare i passi indietro e dire «abbiamo sbagliato» è segno di intelligenza e di prospettiva. Ma perseguire questa strada vuol dire andare a far sbattere questo nostro meraviglioso Paese.

che si sta ritorcendo contro il nostro Paese. Voi non avete deciso una moderata espansione, ma avete programmato uno sforamento senza precedenti e lo avete fatto non per finanziare misure di crescita, ma per iniziare a pagare le cambiali elettorali di questo Governo. Lo avete fatto senza nemmeno scrivere nella manovra quando entreranno in vigore quota 100 e il reddito di cittadinanza, come funzioneranno e quanto costeranno effettivamente. Voi avete innescato con l'Europa non un dialogo intenso e virtuoso - come lei ci ha raccontato oggi - ma uno scontro durissimo e lo avete fatto per puro calcolo elettorale, perché ne volete fare un pezzo della campagna per le europee. E nelle scorse settimane non c'è stato un minuetto tra il Governo italiano e la Commissione europea, ma una sequela di dichiarazioni e di insulti senza precedenti: una cosa mai vista e controproducente, perché ha bloccato qualunque tentativo di cambiare la *governance* della zona euro e di archiviare definitivamente le politiche di austerità che tutti vogliamo superare. Purtroppo per voi avete fatto male i conti, signor Ministro, perché avete sottovalutato la reazione dell'Italia reale, di quel Paese che si alza tutte le mattine per andare a lavorare, che si rimbocca le maniche, che ha da parte qualche euro e vuole evitare che i propri risparmi vengano bruciati dallo *spread.* La fiducia dell'Italia reale è crollata: andate a vedere i dati ISTAT sulla fiducia dei consumatori e delle imprese, che, non a caso, calano da cinque mesi consecutivamente; lo *spread* è andato alle stelle; i tassi per le imprese e le famiglie stanno iniziando ad aumentare. Si sta avverando purtroppo la profezia di Olivier Blanchard, l'ex capo economista del Fondo monetario internazionale: la vostra è nata come una manovra espansiva, ma sta diventando una manovra recessiva che sta portando l'Italia in stagnazione o addirittura indietro. È un capolavoro all'incontrario, signor La sfiducia è talmente cresciuta che l'ultima asta dei BTP è andata semideserta. Guardate che è un campanello d'allarme grave per un Paese che l'anno prossimo deve collocare 400 miliardi di euro di titoli di stato senza l'ombrello protettivo della Banca centrale europea. Il 13 dicembre, signor Ministro, le imprese e gli artigiani del Nord scenderanno in piazza a Milano contro questo Governo ed è la dimostrazione che il giochino della Lega di governo, di potere a Roma e di lotta sul territorio non regge più e anche la parte del Paese che è più impegnata nella competizione economica rigetta la politica di questo Governo. Di fronte a questa malaparata forse vi siete decisi a fare marcia indietro. Io perlomeno ho interpretato così, signor Ministro, le sue parole di oggi. Però lo state facendo, ancora una volta, in modo furbesco e pasticciato, perché perché credo che abbiate paura che il popolo non capisca il «contrordine, compagni», non capisca la marcia indietro rispetto ai roboanti proclami dei Ministri che sul balcone di Palazzo Chigi avevano festeggiato il *deficit* al 2,4. Allora, abbiamo Salvini che da una parte apre, passando dal «tiro dritto» ai decimali che non contano, Di Maio che invece richiude e lei, signor Ministro, che insieme al Presidente del Consiglio, siete - me lo lasci dire - paralizzati da questi veti e da queste posizioni assolutamente divergenti. Signor Ministro, risparmiate agli italiani questo gioco delle tre carte. Non è il momento dei mezzucci, non è il momento dei mezzi passi avanti e dei mezzi passi indietro. Non è il momento dei vertici semiclandestini per non far vedere al popolo la retromarcia. Mettete le carte in tavola: numeri, tabelle ed emendamenti. Cambiate questa manovra e fatelo subito, prima che sia troppo tardi e prima che quel balcone di Palazzo Chigi crolli sotto i vostri piedi, perché prima delle vostre beghe e dei vostri interessi di parte, signor Ministro, ci sono gli italiani e gli interessi dei risparmiatori e dei lavoratori italiani.

Abbiamo ascoltato le sue parole, signor Ministro, e le condividiamo: ne condividiamo i contenuti e gli obiettivi. Le opposizioni vi hanno chiesto di cedere, di mollare, di arrendervi. Noi chiediamo invece al Governo di non fare passi indietro: avete il nostro pieno sostegno. Avete il sostegno della Lega e della maggioranza, quello dei cittadini italiani ed europei che si aspettano un cambiamento, che lo chiedono e lo pretendono. Non c'è alternativa, perché vorrebbe dire arrendersi ad un modello di Europa che spinge alla povertà, all'oppressione e ad un inevitabile declino. Avete la fiducia dei cittadini, andate avanti senza esitazioni. Le attestazioni di apprezzamento quotidiano ai principali esponenti del nostro Governo ne sono una prova. Gli insuccessi elettorali e le contestazioni, anche molto dure, nei confronti degli esponenti politici dei partiti europei tradizionali ne sono una conferma. È paradossale che coloro che oggi giudicano la manovra di bilancio italiana siano esponenti di partiti che sono stati sconfitti e bocciati dai loro elettori. Andate avanti, abbiate coraggio, il popolo è al vostro fianco. Noi crediamo in voi, in un Governo coraggioso che ha l'obiettivo di mettere al centro del modello europeo i popoli e le loro esigenze, non solo i numeri e l'austerità. È ormai dimostrato che le misure restrittive hanno portato al dilagare senza controllo della povertà, della disoccupazione e del disagio sociale, aggravando ulteriormente gli effetti della fase recessiva della nostra economia. L'Italia, dopo la cura Monti e dopo cinque anni di Governi di centrosinistra, resta ancora oggi, al di là delle chiacchiere e delle lezioni che ci vogliono impartire, il fanalino di coda nella crescita della ricchezza tra i Paesi europei. Così non si può andare avanti, sarebbe una follia. È quindi necessario e doveroso cambiare politiche economiche e che questo Governo e questa maggioranza abbiano il coraggio di scegliere una strada diversa, che punti alla crescita, agli investimenti e all'occupazione. I Governi del recente passato hanno ottenuto flessibilità per affinità politiche con i componenti che governano attualmente la Commissione europea

Noi stiamo cambiando le cose: lo stiamo facendo con successo e ne siamo orgogliosi. Nella manovra ci sono precisi impegni per intervenire con misure di finanza pubblica in caso di evidenti difformità rispetto alle previsioni di crescita del Governo. Si ribadisce l'impegno dell'Esecutivo a mantenere sotto controllo l'andamento dei saldi di finanza pubblica, anche attraverso una verifica trimestrale delle spese. Coraggio, quindi, ma anche prudenza e grande senso di responsabilità. Vogliamo il cambiamento, ma nessun salto nel vuoto: non lo vuole nessuno. Vogliamo sfidare i conservatori europei, ma vogliamo che questa sfida abbia successo nell'interesse dei cittadini e delle famiglie italiane. Prosegua quindi il dialogo con gli attuali vertici europei, ma senza recedere di un passo rispetto ai princìpi e alle determinazioni che hanno ispirato la formazione di questo Governo. Nella consapevolezza di rappresentare la maggioranza degli italiani, chiediamo rispetto da parte della Commissione europea, anzi, lo pretendiamo. Non possiamo e non vogliamo fare passi indietro rispetto alla strada tracciata. Gli obiettivi della legge bilancio sono chiari e li condividiamo: investimenti pubblici e privati per rilanciare l'economia; lotta alla povertà e redistribuzione del reddito; attenzione ai nostri giovani che cercano lavoro e che vogliono costruirsi un futuro in Italia; rispetto per chi ha lavorato una vita e ha diritto a una pensione dignitosa; tutela dei diritti dei risparmiatori truffati e traditi dai Governi precedenti; un fisco più equo che stimoli i consumi e la crescita. Il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione non è disposto a sostenere l'azione di un Governo che non abbia coraggio e non punti al cambiamento. Siamo pienamente consapevoli di aver intrapreso un percorso difficile, ma non abbiamo alcuna intenzione di fermarci, tanto meno di tornare indietro. La continuità con le politiche del passato porterebbe ad un sicuro insuccesso, al fallimento non tanto di un Governo, del nostro Governo, ma dell'intero Paese. Rappresentiamo la speranza della maggioranza degli italiani e non dobbiamo mai scordarcelo: andremo avanti accettando ogni sfida, con senso di responsabilità, coraggio e determinazione.

ha parlato di dialogo virtuoso con la Commissione europea e di clima di fiducia, che lei ritiene possa cambiare, e dunque di darle credito su questo aspetto. Preliminarmente, però, le pongo una domanda: è la sua opinione, questa sul dialogo virtuoso e sul clima di fiducia?

quando parliamo in queste sedi e quando lei parla nelle sedi europee, è che il clima è completamente diverso dal dibattito politico e dai due *leader* di questa maggioranza. Vede, signor Ministro,

quest'azione macroeconomica di tipo negativo ci pone di fronte al rischio reale che chi sta bene starà sempre meglio e chi sta male starà sempre peggio, con un piccolo problema, ossia un punto di rottura che veramente ci preoccupa. Nella società civile, permettetemi questa breve citazione personale, sono un imprenditore e vengo dal Nord, anzi da quel Nord-Est che, fino a qualche anno fa, era considerato la locomotiva del nostro Paese

inserito anche un rallentamento economico italiano ed europeo che nel terzo trimestre del 2018 ha confermato tale tendenza negativa, impone scelte forti.

Lei mi insegna e ha insegnato, come del resto insegnano tutti, che con la spesa corrente non si va a modificare il PIL. Con l'indebitamento fine a se stesso non si modificano i nostri saldi finali.

qualche collega ha parlato di cifre, i piccoli e medi imprenditori sono artigiani, imprenditori agricoli, coltivatori diretti o falegnami; ebbene, cosa volete che ne sappiano di fattura elettronica? Li stiamo caricando di un costo ulteriore. Tornando alla manovra: perché

Volete un Paese in cui ci sia gente che lavora e gente che consuma; noi vogliamo aiutare quella parte del Paese che lavora, che produce, che ha permesso al nostro Paese di uscire da crisi ben più gravi di quella attuale. Signor Ministro, personalmente ho molta fiducia in lei: si faccia sentire, batta i pugni non solo a Bruxelles, ma anche a Palazzo Chigi. Si faccia ascoltare. Buon lavoro.

signor Ministro, condividiamo pienamente la sua analisi e la sua ricostruzione dei fatti. L'Europa ci ha fatto un richiamo, facendo il primo passo per un'eventuale procedura di infrazione per debito eccessivo. Sicuramente le istituzioni europee preposte a questi interventi si intendono di numeri, ma mi pare di capire che abbiano anche una cultura classica perché la lettera con cui, sostanzialmente, si contesta la manovra economica mi ha ricordato la famosa favola di Fedro del lupo e dell'agnello, che bevono allo stesso ruscello, ma il lupo, che è a monte, accusa l'agnello, che è a una certa distanza ed è a valle, di intorbidire l'acqua. infatti, l'Unione europea fonda la sua contestazione non sulla violazione del rapporto *deficit-*PIL del 3 per cento, visto che la manovra di questo Governo lo prevede al 2,4, ma contesta che il debito scenderà poco nel 2019,

Il documento dice testualmente: «Sulla base dei dati notificati e delle previsioni dell'autunno 2018 della Commissione, l'Italia non ha rispettato il parametro di riduzione del debito nel 2016

«complessivamente, la mancanza di conformità dell'Italia con il parametro di riduzione del debito nel 2017 fornisce la prova dell'esistenza *prima facie* di un disavanzo eccessivo ai sensi del patto di stabilità e crescita, considerando tutti i fattori come di seguito esposti. Inoltre, in base ai piani governativi e alle previsioni dell'autunno 2018 della Commissione, l'Italia non dovrebbe rispettare il parametro di riduzione del debito nel 2018 o nel 2019». Come sappiamo, i Trattati prevedono che i debiti dei Paesi dell'Unione europea debbano tendere al 60 per cento, ma tanti Paesi sono lontani da questa soglia e si prevede che per il 2019 il debito medio per i Paesi dell'Unione europea sia dell'85

Come si è detto, proprio sul debito eccessivo degli anni 2016 e 2017 si basa la contestazione odierna dell'Unione europea e l'eventuale apertura della procedura di infrazione.

mi verrebbe da dire che le colpe dei padri ora devono ricadere sui figli, secondo l'Unione europea. La verità è tutta al contrario rispetto a quanto ci dice l'Europa: è stata proprio l'austerità insensata che è stata imposta dai tecnocrati dell'Unione europea a far esplodere Il debito pubblico è aumentato di circa il 30 per cento in dieci anni proprio applicando le politiche dell'Unione europea. europea. Noi amiamo il nostro Paese, difenderemo i suoi interessi con tutte le nostre forze e faremo valere gli interessi dei cittadini italiani davanti a qualsiasi organismo europeo. Faremo prevalere il buon senso e le buone pratiche di governo. *(Applausi

di tipo accademico che mi sono venute e che mi hanno fatto sorridere, ma ritengo di non farlo, perché non credo che sia di interesse del Senato.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, che dire? Lei ha fatto un intervento parlando di necessità di equilibrio, dicendo che il Parlamento e il Governo, con responsabilità, devono tenere conto degli equilibri complessivi. Ha detto che bisogna mantenere un equilibrio tra la spesa e gli investimenti, che bisogna dialogare e avere un rapporto costruttivo con l'Europa. Ora, la mia domanda è:

Che il ciclo non fosse positivo era chiaro; che tutti gli osservatori internazionali e nazionali sostenessero che la vostra previsione di crescita non fosse credibile era chiaro; che cos'è successo? L'altra domanda, cui non avrò risposta, è questa: forse vi siete resi conto

capire così? Ormai la verità sta in poco posto, al di là di tutti i numeri. Lo *spread* produce un rischio di *credit crunch* per le imprese, un danno per i risparmiatori e un danno per

lei qui ha parlato a nome del Governo oppure no? Non vorrei che il tentativo che ora state facendo sia sostanzialmente questo: allunghiamo i tempi, aspettiamo le elezioni europee e le correzioni si faranno dopo.

bisogna spostare le spese in *deficit* sugli investimenti, come ha detto lei. In secondo luogo, bisogna che questi investimenti

dovete cambiare la legge di bilancio e produrre uno sforzo per mettere in condizione gli enti locali, le Regioni e il sistema della pubblica amministrazione di realizzare investimenti con un grande piano sulle opere per la messa in sicurezza del territorio e un piano di assunzioni. Ciò può consentire di invertire la

Il vice presidente Salvini dice che la manovra non c'è finché non è approvata in Parlamento. Ci dobbiamo attendere che in terza lettura farete le modifiche per arrivare fino alle elezioni europee oppure avrete il coraggio di dire che avete fatto un errore grave nel costruire una manovra senza una strategia chiara e un confronto rivolto insulti gravi alla Commissione che non porteranno nulla a questo Paese, se non danni per i cittadini e le imprese?

Signor Ministro, abbiamo ascoltato con interesse le sue parole, che purtroppo non ci convincono. Tuttavia, le riconosciamo uno stile e una compostezza che nel rapporto con l'Unione europea ci piacerebbe vedere anche in molti dei suoi colleghi. Oggi l'Unione europea chiede all'Italia responsabilità sulla manovra di bilancio e sulla gestione complessiva dei nostri conti, perché, come ha ricordato il Presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, i Paesi con un alto debito sono vulnerabili. Ci vuole quindi prudenza, soprattutto quando la situazione dell'economia internazionale vede diverse minacce. E poi c'è anche un tema di rispetto delle regole: altri Paesi lo seguono, perché per l'Italia non dovrebbe valere? Signor Ministro, noi crediamo che questo Governo si dovrà impegnare per ritrovare considerazione in ambito comunitario. Questo atteggiamento di scontro, unitamente a una manovra basata su nuovo debito, ci ha isolati anche all'interno dei cosiddetti amici sovranisti di questo Governo,

Lo *spread* è passato da 130 a quota 300 e, come lei ha ammesso alla Camera dei deputati, la principale conseguenza sarà l'aumento del costo dei nuovi mutui e la difficoltà di accesso al credito per le imprese. Banca d'Italia ha calcolato che, con questa vostra politica, gli interessi sul nostro debito sono aumentati di 1,5 miliardi quest'anno e aumenteranno di ben 14 miliardi per i prossimi due anni. Tutta questa situazione sta generando incertezza e paura nei risparmiatori. Non a caso, la settimana scorsa, con la vendita dei BTP nazionali, sono stati prestati dai risparmiatori allo Stato appena 2,3 miliardi di euro, mentre nel maggio Questi dati la dicono lunga sulla vostra strategia economica. Oggi annunciate di voler rivedere al ribasso le cifre della manovra. Tuttavia, a mio avviso, la questione non è di decimali, in quanto legata all'impostazione stessa della manovra, perché non basterà spostare alcuni miliardi sulla crescita e sullo sviluppo se prima non si mettono in campo riforme significative, in grado di dare senso anche a misure come il reddito di cittadinanza. Siccome voi parlate sempre di un piano che punta al lungo termine e alla durata dell'intera legislatura, in questo primo anno avreste dovuto aggredire la burocrazia, procedere con una riforma della giustizia, semplificare l'accesso al credito e tagliare le tante leggi inutili di cui

Purtroppo, invece, voi introducete oggi il reddito di cittadinanza e lo fate in un Paese in cui i centri per l'impiego sono in una condizione disperata, senza *computer*, personale adeguato e la messa in rete di tutte le informazioni. Fate tutto questo in un Paese dove ancora forte è il lavoro in nero e, prima, e, prima, ci sarebbe voluta una forte iniziativa per contrastarlo. Dubito pertanto che questa saprà essere una misura attiva per il lavoro e credo che porterà solamente nuovo debito pubblico, senza aiutare la gente a migliorare le proprie condizioni. Per questo motivo, l'invito che facciamo è a rivedere il più possibile una manovra che sarà deleteria per i nostri conti pubblici e non porterà abbastanza benefici alla crescita. Tutti gli organismi internazionali dicono che l'economia italiana frenerà e non si capisce come mai sia solo il Governo a fare stime così diverse da tutti gli altri. Google Trends ci dice che la parola «*spread*» ha superato nelle ricerche sulla rete le espressioni «reddito di cittadinanza» e «*flat tax*», diventando la più importante delle ultime settimane. L'incertezza e il timore che le cose vadano peggio stanno prendendo il posto delle attese per le promesse elettorali. Ascoltate allora il consiglio di Tsipras, che sa di cosa parla, e abbandonate una manovra che, nel suo insieme, poggia su una visione di corto respiro che non guarda al futuro. L'oggi al posto del domani è stato il vizio peggiore della politica italiana. Per questo si continui il dialogo con l'Europa e si imbocchi con convinzione la strada della responsabilità anche nei confronti delle future generazioni e dell'interesse generale.

Grazie,

la maggioranza e i Ministri sono impegnati in un duro braccio di ferro con l'Unione europea. Sia ben chiaro che anche noi riteniamo che l'attuale

degli effetti della globalizzazione, della perdita di potere d'acquisto delle nostre famiglie, della sofferenza di interi ceti sociali. Potremmo parlare anche in questa sede dello *spread* e della sua capacità di riflettere esattamente e correttamente lo stato di salute di un'economia, ma il tempo è poco. Vede, signor Ministro, se la guerra che voi avete intentato all'Unione europea fosse costruita intorno al programma che il centrodestra ha presentato alle elezioni, noi saremmo al vostro fianco in questa battaglia. voi aveste presentato alla Commissione europea un testo che prevedesse il taglio forte e deciso delle tasse nei confronti dei cittadini, delle imprese e delle famiglie, noi saremmo al vostro fianco. Se in questa manovra ci fosse una traccia della *flat tax*, se in questa manovra ci fosse un'ombra almeno di quegli investimenti ad alto moltiplicatore, ad alto valore aggiunto di cui ha parlato molto spesso il ministro Toninelli, noi saremmo al vostro fianco. Il problema è che di tutto questo non c'è assolutamente nulla, Ministro. Questa manovra, purtroppo, duole dirlo, è concentrata su una sola esigenza primaria, direi assorbente rispetto a tutte le altre esigenze: quella di garantire dieci miliardi di spesa corrente al MoVimento 5 Stelle, fatto in debito per pagare la promessa elettorale del reddito di cittadinanza. *(Applausi dal Gruppo FdI)*. Altro non c'è in questa manovra. È tutto qua, purtroppo, il senso della manovra finanziaria e dello scontro che abbiamo con Bruxelles. Come questo possa stimolare la crescita per noi rimane Grazie, e poveri noi - la fine della povertà, ha consentito ad un Ministro della Repubblica di annunciare la stampa di cinque, forse sei milioni di tessere prepagate da distribuire in vigilia di campagna elettorale (anche questa è una scena che questo Paese forse non meritava) e molte altre occasioni di propaganda. Adesso, Ministro, lei e altri autorevoli esponenti del Governo comunicate che la rigidità rispetto al *deficit* fissato al 2,4 per cento non è più tale. Qualcuno dice che si tratta di numerini. Ebbene proprio numerini non sono. Lei lo sa meglio di me, Ministro, che un decimo di di PIL vale 1,7 miliardi e due decimi sono 3,4 miliardi, che rischiano di avere effetti anche sulla credibilità della crescita del PIL che voi avete messo nero su bianco nel documento

più ha destato scalpore riguarda una trasmissione televisiva di cui si è molto parlato in questi giorni e che ha riguardato le attività familiari di un Ministro, di cui a me però personalmente non interessa assolutamente nulla perché penso che la politica si debba fare su altri piani si possa salire sul *ring* della politica e battersi anche forte, ma rispettando alcune regole di civiltà. Ma questo, del resto, è il precipitato di iniziative politiche che hanno delle responsabilità molto precise. A parte questo, quello che mi ha molto colpito di quella indagine giornalistica, signor Ministro, è Ministro, è la registrazione precisa della pervasività del lavoro nero nel nostro Paese e ho pensato che quel lavoratore oggi sarebbe sicuramente un percettore di reddito di cittadinanza e che, come lui, molte persone che magari al Sud hanno un piccolo impiego con contratti *part time* o di apprendistato rinunceranno a lavorare per ottenere il reddito di cittadinanza. Ho pensato che molte persone rinunceranno a cercare un lavoro per ottenere il reddito di cittadinanza e è triste quel Paese che incentra una battaglia 18 contro 1 soltanto per questo motivo. Alla fine voi ci portate a discutere di una manovra finanziaria che ha due grandi poli di riferimento: quota 100 e reddito di cittadinanza. Qui abbiamo la rappresentazione di un Paese in cui c'è un pezzo di Paese che non vede l'ora, legittimamente, di smettere di lavorare e un pezzo di Paese di cinque-sei milioni di persone che non vuole nemmeno iniziare a lavorare. In mezzo, però, c'è il Paese reale, di cui questa manovra non parla, di cui non si occupa più nessuno, i ceti produttivi, le persone che si alzano presto la mattina per andare a lavorare, gli operai, gli impiegati, gli agricoltori. Tutto questo mondo è completamente dissolto perché si parla soltanto di interventi assistenziali e improduttivi, certamente molto efficaci dal punto di vista elettorale, ma la domanda è se siano efficaci anche per la tenuta internazionale di questo Paese. Noi abbiamo molti dubbi. Avete privilegiato la politica dell'assistenza del bisogno e avete completamente dimenticato la politica del merito. Ci sono 100.000 giovani che ogni anno lasciano questo Paese e che non vogliono il vostro reddito di cittadinanza, non vogliono l'elemosina di Stato, non vogliono il metadone di Stato, vogliono un Governo che consenta loro di dimostrare che i sacrifici che hanno fatto valevano qualcosa, vogliono la dignità che nasce dal lavoro e in questa manovra finanziaria purtroppo di questo non c'è traccia. C'è molto che riguarda la distribuzione del reddito, ma non c'è nulla rispetto a chi il reddito lo deve creare creando ricchezza. C'è molto legato a domani, a dopodomani o al 28 maggio, ma nulla rispetto a quello che potrà accadere dopo. Lei, signor Ministro, a cui riconosciamo serietà, sicuramente sente su di sé le responsabilità che derivano da fatti molto precisi e molto inquietanti: il fallimento della gara dei buoni poliennali del tesoro, il rallentamento dell'economia, il rallentamento dei consumi, il rallentamento dell'economia internazionale. Le chiedo se onestamente lei pensa che quanto ci è venuto a raccontare oggi sia la soluzione per questo Paese. Io ritengo proprio di no. Signor Ministro, lei ha l'incarico da parte della sua maggioranza, ma anche del Parlamento e di tutto il Paese, di andare a Bruxelles non per chiedere per l'Italia una deroga, la possibilità di farla franca, ma semplicemente lo stesso trattamento che ricevono tutti gli altri Stati, la stessa dignità, la stessa la stessa responsabilità. Se lei farà questo, ancora una volta, come sempre, noi saremo al fianco dell'Italia, del Paese, della Nazione, se viceversa farà quanto purtroppo temiamo faccia, ci troverà coerentemente ancora una volta all'opposizione.

colleghi, abbiamo ascoltato con grande attenzione la sua relazione e le confesso che avremmo preferito ascoltare parole importanti anche nella sua replica. Purtroppo, il suo silenzio è entrato in sintonia perfino con la risoluzione presentata dalla maggioranza, che mi auguro sia un'assenza cartacea, più che un'assenza di proposte, di idee e di programmi per il futuro di questo Paese. Abbiamo ascoltato con interesse la sua riflessione iniziale sottolineando - e lo voglio dire immediatamente - che la necessaria riapertura di una relazione con l'Europa è sicuramente un passo in avanti, anche se avviene in maniera tardiva,

e più in generale ancora con la presentazione di una manovra che - non dobbiamo dimenticarlo, signor Ministro - si sta discutendo alla Camera dei deputati e probabilmente sarà molto diversa rispetto a quella che verrà approvata, ma ancora oggi non è dato capire quali saranno i nuovi saldi, le nuove prospettive, le nuove proposte che riallineeranno il contesto italiano al contesto necessario per rigenerare stabilità, crescita, affidabilità e serietà nella gestione dei conti pubblici.

il cuore fondamentale delle parole che lei ha anche introdotto, Ministro (responsabilità nazionale, esigenza di sostenere gli investimenti per il futuro del Paese) è a nostro avviso completamente in contrasto con il contratto di Governo; il contratto di Governo; un contratto che viene venduto e contrabbandato come un investimento importante per il futuro del Paese, ma che in realtà nasconde al suo interno un pericoloso e insidioso ritorno al passato, a politiche che usano il debito per incrementare la spesa, fanno diventare i sussidi, le mance, i condoni, elementi strutturali che sostituiscono gli enormi investimenti necessari nell'istruzione, nella salute, nell'università e nella ricerca. contratto è un gigantesco ritorno al passato, al cui interno, peraltro, insiste un equivoco strutturale che ritengo inaccettabile: continuare a fare opposizione al passato senza garantire nessuna proposta per il futuro e per lo sviluppo economico di questo Paese. questo è un elemento artificiale che può essere utile alle elezioni, ma un Governo non nasce esclusivamente per piegare le proprie azioni alle elezioni. Nasce, e apre un ciclo, se è in grado di guardare alle generazioni, al futuro di questo Paese, allo sviluppo economico dello stesso, ai suoi fondamentali elementi di investimento. È un pericoloso ritorno al passato per queste ragioni: perché dovete sempre e comunque ricercare nemici per un consenso elettorale. È stato così con l'Europa, ma è così anche in Italia: si cerca inevitabilmente il nemico, che in questo caso individuate in chi ha governato il Paese negli anni precedenti, peraltro senza mai tener conto delle azioni che ci hanno portato a garantire un recupero della crescita, un recupero di una fase difficile che l'economia globale ha attraversato, invertendo i segni e trasformandoli da negativi in positivi, nel lavoro, nell'occupazione e anche nella riduzione della pressione fiscale e nel rilancio degli investimenti. Ancora più grave è che annunciate l'accusa usando i pilastri fondamentali del Governo precedente. Diciamocelo con chiarezza: i due fondi che stanno paralizzando la manovra sono il reddito di cittadinanza e quota 100. Sarebbe stato molto più semplice se non ci fosse stata la volontà di fare opposizione al passato rafforzando il reddito di inclusione, la prima misura universale che il Governo precedente aveva introdotto dal Gruppo PD)*. Forse non eravamo riusciti a contrastarla per intero, ma quella è la prima misura universale sulla quale poggia, peraltro, la vostra propaganda su un reddito di cittadinanza che che introduce una misura assistenziale, non utile a contrastare povertà, solitudine e indifferenza, ma utile a mantenere un impegno elettorale nei confronti degli elettori,

perché avete cancellato le strutture di missione utili a generare un nuovo piano nazionale per il contrasto del dissesto idrogeologico. L'Italia ha bisogno di un piano di manutenzione straordinaria, e non lo si fa attraverso una centrale unica né con Sviluppo Italia. Lo si fa se si ridanno ai Comuni le condizioni fondamentali per poter ripartire negli investimenti nella dimensione territoriale. *(Applausi un enorme processo di cambiamento, ma in realtà state producendo un ritorno al passato pericoloso, per i contribuenti, per le famiglie, ma soprattutto dannoso per lo sviluppo economico e sociale. State riuscendo a fare il contrario di quanto dovremmo fare se vogliamo avere a cuore l'Italia; quell'Italia che volete rappresentare a parole, ma che nei fatti non riuscite a rappresentare perché mancano le misure fondamentali: manca il cuore di un'idea del futuro del Paese. Per questo voteremo la nostra risoluzione, che abbiamo rappresentato per dare voce alle famiglie e alle imprese italiane che cominciano anche in questi giorni a non trovare nell'azione del Governo le basi fondamentali per costruire sviluppo e crescita.

il dibattito odierno ci ha consegnato l'immagine piuttosto nitida delle idee e dei valori che si misurano sotto la superficie di una contesa solo apparentemente incardinata su numeri e parametri. Siamo una forza parlamentare responsabile, che conosce bene l'importanza degli obblighi internazionali e l'esigenza di qualificare il Paese nella percezione dei mercati in termini di affidabilità, ma non possiamo né vogliamo rinunciare al ruolo proprio, nobile e alto della politica. Non si governa l'Italia e nemmeno l'Europa contro gli italiani e contro gli europei. Se le regole che si pretende e ci si ostina ad applicare non funzionano, è compito della politica metterle in discussione e, se necessario, cambiarle. Veniamo da due lustri di misure restrittive. I loro effetti li subiscono già oggi - non c'è bisogno di attendere il futuro - sulla propria pelle milioni di italiani sprofondati in stato di povertà; si manifestano in un crescente disagio sociale, nell'aumento della disoccupazione, in una complessiva perdita di competitività del Paese. Questa maggioranza ha scelto una netta inversione di rotta rispetto al passato ed ai suoi esiti. Riteniamo che occorra una politica economica declinata in misure anticicliche capaci di contenere gli effetti della fase recessiva e rilanciare la crescita, partendo da una ripresa significativa della domanda interna. Non sono valutazioni estemporanee, ma trovano conferma precisa e scientifica nelle elaborazioni di economisti come il premio Nobel Paul Krugman o di Richard Koo, il primo studioso della crisi asiatica della fine del ventesimo Tutti concordano, nel solco della lezione keynesiana, che nelle congiunture come quella attuale di dimensione sistemica si debbano adottare politiche espansive. Lo stesso Fondo monetario internazionale ha dovuto rivedere le proprie posizioni dinanzi alla spirale recessiva alimentata dall'*austerity*, ammettendo che perseverare nell'utilizzo di moltiplicatori calcolati nel periodo precrisi potrebbe provocare effetti ancora più negativi. La manovra proposta dal Governo va proprio in questo senso, offrendo uno stimolo all'attività economica e alla domanda privata finalizzato a realizzare un più alto livello del PIL nominale, così da ridurre nel triennio il rapporto debito-PIL operando anche sul denominatore. Il *deficit* programmatico per il 2019 al 2,4 per cento contiene peraltro - e nessuno lo ha citato - la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia relative all'incremento delle aliquote IVA e delle accise sui carburanti, sulle quali tutte le forze presenti in Parlamento avevano assunto precisi impegni con i cittadini italiani. Signor Ministro, l'impegno del Governo a mantenere sotto controllo l'andamento dei saldi di finanza pubblica, anche attraverso un controllo trimestrale delle spese, rappresenta la chiara volontà di perseguire una gestione dei conti più responsabile che in passato e una buona base di partenza per aprire un confronto ampio e aperto con le istituzioni europee. confronto non può però rinunciare alla nostra *Weltanschauung*, alla nostra visione del mondo, della quale siamo latori. È l'uomo, il cittadino al centro; L'economia e la finanza devono tornare a essere strumenti in mano all'uomo per regolare e governare le risorse. Non possiamo più accettare che siano i numeri e i parametri della finanza e dei mercati a determinare le vite, la povertà e l'infelicità della gente. Senza scomodare la morale benthamiana, noi siamo davvero convinti che il valore della felicità pubblica sia quantificabile e dunque possa essere assunto come criterio dell'agire. Bentham formulò un'algebra morale, cioè un calcolo quantitativo delle conseguenze dell'agire pubblico in termini di felicità collettiva prodotta. Noi vorremmo un'Europa attenta agli effetti delle politiche pubbliche, anche di bilancio, sulla vita dei cittadini e, nella consapevolezza della perfettibilità di ogni scelta, ribadiamo il nostro sostegno all'azione del Governo perché massimizzi l'interesse e la felicità degli italiani. Per tutte queste ragioni, a nome del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione,

un concetto che accomuna tutto il Gruppo Forza Italia. Signor Ministro, noi tifiamo per l'Italia, noi tifiamo per il nostro Paese, noi siamo accanto ai nostri concittadini: questo bisogna metterselo chiaro e tondo in testa. Non è che qui, se uno intende criticare la vostra manovra, è come se si ponesse in netto contrasto con i nostri concittadini.

che ha l'onere di governare questo Paese. Pertanto, la sua prosopopea, che ha utilizzato nella replica, la vorrei archiviare come una caduta di stile. Non voglio utilizzare le parole del sottosegretario Castelli, che ha affermato semplicemente: «Lei lo dice». Abbiamo un altro stile. Noi rispettiamo le persone che si sono formate. Spero per lei, non per noi, che non cada più, che non abbia più questa cessione di stile. Signor Ministro, che sia chiaro: a noi non mette paura la vostra discussione, anche accesa e virulenta, con l'Europa. Noi in tempi non sospetti abbiamo detto che questa Europa non ci convince; lo abbiamo detto nel 2005 - lei non se lo ricorderà - in occasione dei Trattati dell'Unione.

Paesi su diciannove sono critici verso questa manovra; non può essere un complotto, non può essere archiviato come un complotto internazionale. Come le dicevo, non ci mette paura l'Europa e non ci mette paura neanche lo *spread*.

Signor Ministro, don Luigi Sturzo diceva che una manovra non si inventa, ma si vive. Noi temiamo che qui rischiamo di non sopravvivere In quest'Aula c'è una parte importante della compagine governativa che fa riferimento alla cultura dei sovranisti, questa nuova dottrina. Allora prendiamola in esame. La dottrina dei sovranisti è: prima l'io nazionale e poi il noi europei.

C'è il reddito di cittadinanza, e lo voglio dire a chiare lettere: noi non contestiamo il reddito cittadinanza, che è certamente un provvedimento di inclusione sociale e di giustizia sociale. Noi contestiamo le modalità e la tempistica con cui lo state attuando. Prima avremmo dovuto occuparci del taglio del cuneo fiscale, di rilanciare l'economia, di rilanciare l'occupazione, di aiutare le imprese; poi avremmo potuto studiare questo strumento. Lei lo sa meglio di me, perché abbiamo svolto diverse audizioni: lo stipendio medio di un ragazzo sotto i trentacinque anni appena assunto al Nord è di 930 euro, lo stipendio medio dello stesso ragazzo assunto al Sud è di 740 euro netti al mese. Come fa a dire il vice presidente Di Maio che questo provvedimento avrà un effetto positivo sull'occupazione? È un'affermazione del tutto destituita di fondamento. FI-BP)*. Caro Ministro, non posso non aprire una parentesi sul lavoro nero in questo Paese: lo chiede l'attualità. Lei sa meglio di me che la CGIA di Mestre con uno studio ha affermato che in questo Paese ben 37 miliardi di euro non vanno nel fisco e non vanno nelle casse dello Stato a causa del lavoro nero.

non chiedeteci di abdicare e rinunciare ai valori e alle idee che abbiamo inserito nel nostro programma comune, quello che abbiamo presentato ai nostri cittadini. Non possiamo farlo e non possiamo abdicare a quelle idee, perché quel programma elettorale non solo contiene idee e progetti di natura economica, ma contiene un patto che abbiamo scritto con i nostri concittadini e quel patto si fonda sul nostro DNA culturale e valoriale. Noi a questo non intendiamo rinunciare.

se l'Europa è destabilizzata, non è per colpa della manovra economica e finanziaria degli italiani. Se l'Europa è destabilizzata è perché ha venduto la propria anima comunitaria ai mercati della finanza! Come fate a

impoveriamo questo Paese. Io vi vorrei invitare ad accompagnarmi a casa stasera e a fare il Lungotevere e passare attraverso il colonnato di via della Conciliazione.

Ci sono 5 milioni di italiani che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Ci sono famiglie che fanno fatica a sopravvivere. Ci sono aziende che stanno chiudendo. Ci sono persone che stanno gridando la loro disperazione e voi continuate a parlare dai Gruppi FI-BP e PD)*. Noi dobbiamo cercare di restare uniti e dobbiamo cercare di vedere le cose da una prospettiva che non può essere quella della logica della contrapposizione ideologica, soprattutto quando poi apriamo il fronte che ci vede in questo momento in anteposizione con l'Europa.

che con 300 miliardi di debito pubblico in sette anni solo uno Stato suicida avrebbe potuto continuare in quella direzione. Eppure ci avevano detto che il *jobs act* avrebbe fatto volare l'economia; ci avevano detto che l'articolo 18 era il freno alla produttività delle nostre aziende e che, se avessimo tolto l'articolo 18, le nostre aziende sarebbero volate e sarebbero diventate finalmente competitive!

che la globalizzazione e il neoliberismo sono ormai implosi, perché non facevano circolare le idee, ma le merci.

dove la democrazia, come noi la intendiamo, vuol dire necessariamente una prospettiva di sviluppo sociale e di giustizia da attivarsi nella libertà. *(Commenti dai queste sono le aspirazioni cui legittimamente deve tendere un popolo, non importa se sia il popolo italiano o francese. Queste sono le idee che devono dare forza all'Europa, devono fortificare quel senso di unità che in questo momento realmente difetta in Europa. Certo, stiamo stiamo vivendo e ci accingiamo a vivere i difficili momenti della ricostruzione di un Paese, perché la povertà e l'avvilimento dovranno naturalmente essere sostituiti da questa feroce volontà di rinnovarsi e rinascere. Sono difficili i momenti come questo e come quelli che ci attendono nei prossimi mesi, ma non possiamo fare finta di non sapere che ci sono giovani che in questo momento devono lasciare le proprie case per emigrare all'estero e trovare lavoro. Non possiamo far finta di non sapere che i giovani più coraggiosi, quelli che restano qui, vengono presi al gancio del precariato a vita e del sottopagamento dei lavoratori, a nero.

Non buttiamola ogni volta in confusione, perché mi sembra che la cosa sia sufficientemente grave per poter essere discussa e votata entro i termini temporali che sono stati da voi richiesti. VOCE DAL GRUPPO PD.

prende il disoccupato cronico e, poiché è figlio di un mestiere che nessuno più chiede, lo accompagna verso una nuova formazione professionale, lì dove può avere una speranza

Senatori, c'è un collega che ha preso la parola per un voto in dissenso e credo che abbia assolutamente la dignità e il diritto per poterlo concludere.

Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione le comunicazioni del Ministro, ho rilevato con interesse gli elementi di novità rispetto alle precedenti posizioni non del ministro Tria, ma del Governo. Considero tali elementi di novità non già come segni di cedimento alle osservazioni dell'Unione europea o alle pressioni dei mercati, bensì come segno di un'evoluzione verso un esercizio più responsabile, più realistico e più proficuo della sovranità

la politica migliore per proteggere i più deboli e i più poveri in una società è quella di impedire alti tassi di interesse. con riferimento specifico alle comunicazioni rese oggi dal Ministro dell'economia e delle finanze sulle decisioni in materia di bilancio, il mio voto sarà favorevole.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 Senatore Marcucci, non ritorni sull'episodio di prima, perché prima di aver letto il Resoconto stenografico, non posso assumere alcuna decisione. Le tolgo la parola se il suo

presiedere i lavori nelle prossime ore. Quindi, voglio lasciare subito agli atti che il Resoconto stenografico va esattamente nella direzione della nostra protesta e che gradiremmo, all'arrivo del Presidente del Senato, che sia attivato l'atto di censura a norma dell'articolo 67.

Vi è da dire, però - e lo faccio con grande serenità e veramente con l'intenzione di rasserenare i toni - che in quest'Aula si sono sentite più volte,

con maggiore o minore intenzione nel proferirle - si pronunciano e non mi sembra che possano esulare, Presidente (al di là di una valutazione), da quello che è il normale esercizio dell'attività e delle prerogative del collega.

Su questa riforma è intervenuta una sentenza del Consiglio di Stato, che ha rimandato il testo in Europa e si attende, quindi, un verdetto della Corte europea. Ci troviamo, dunque, di fronte a un caso tipico di conflitto tra i poteri: da una parte, c'è una legge che dice ad alcune banche popolari che devono indire le assemblee per trasformarsi in SpA dall'altra, c'è una sentenza del Consiglio di Stato che dice loro che devono attendere, perché la Corte europea devi dire se quella riforma è legittima o meno su alcuni aspetti importanti che riguardano gli azionisti di quella banca. banca. In un caso del genere, quindi, una proroga è in qualche modo obbligatoria. Il mio emendamento chiedeva una proroga di due anni, ritenendo questi tempi fisiologici attraverso i quali ci potrà essere un'espressione certa da parte dell'Europa e anche un certo lasso di tempo per metter mano - io spero - a quel problema del credito di prossimità che la che la riforma delle popolari e delle banche di credito cooperativo nella scorsa legislatura ha posto in termini drammatici, soprattutto per quel che riguarda i territori meridionali. ha ritenuto di intervenire con un emendamento identico, che fissa la proroga di un anno al al 2019 e non al 2020. Per questo, Presidente, le avrei chiesto e le chiedo una riformulazione del mio emendamento, ponendo «2019» al posto di «2020», in modo tale che l'emendamento diventa identico a quello della Commissione e possa essere votato insieme a quello della Commissione ora che lei lo ha messo ai voti.

per il terremoto del 2008 dell'Emilia-Romagna. Con tutti i condoni che si stanno facendo, non si capisce perché, laddove c'è ancora una dichiarata

gli agriturismi non vengano tassati in quanto sono un'attività a sostegno dell'attività agricola. Nello stesso tempo, ai fini fiscali chiediamo di considerare equiparati ai coltivatori diretti iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale gli appartenenti ai rispettivi nuclei famigliari iscritti nella medesima gestione. Riteniamo che questi tre interventi abbiano un senso e soprattutto

C'è una parte minoritaria della norma che affronta la questione fiscale delle zone economiche speciali, ma la parte prevalente interviene in materia di trasportistica che è di prevalente competenza delle Regioni e per cui ci vuole l'intesa con le Regioni. Lo dico non solo a memoria documentale, ma perché stiamo invadendo l'autonomia

dei beni relativi alle reti di accesso appartenenti a diversi operatori in un soggetto giuridico non verticalmente integrato e *wholesale,*» - chiedo al Governo di indicare in italiano

vuol dire che stiamo parlando di scorporo della rete Telecom; vuol dire che si fa un'unica società - un unico veicolo pubblico-privato, suppongo

Penso sia un problema sul quale valga la pena che quantomeno la Commissione industria faccia un approfondimento. Mi dicono che in Commissione bilancio non se ne sia parlato: l'emendamento è passato come se fosse una proposta qualunque.

si sta parlando della più grande infrastruttura digitale che il nostro Paese si appresta a varare. Si parla di un impegno che uno dei Governi precedenti, per la precisione nel 2015, prese prese nei confronti dell'Europa: l'impegno a digitalizzare il Paese. Digitalizzare il Paese vuol dire raggiungere l'85 per cento della popolazione italiana con una infrastruttura digitale di 100 megabit;

Paese. Io non sono contrario al fatto che una volta tanto si risolva in sede normativa un problema di questo rilievo; mi sorprende però che lo si risolva con un emendamento al decreto fiscale; mi sorprende che si faccia un emendamento di questo tipo senza fare i conti con quello che accadrà. Un esempio che vale per tutti: TIM oggi ha debiti per 28 miliardi, ha un EBITDA di 6 miliardi all'anno (quindi teoricamente sarebbe in grado di diminuire il debito), vanta decine e decine di migliaia di collaboratori. Se quanto è previsto nell'emendamento si dovesse verificare, vuol dire che TIM dovrebbe rinunciare a una parte del debito a favore della rete che si va a costruire, vuol dire che 30.000 dipendenti di TIM dovrebbero

è un problema così enorme che mi sembra francamente riduttivo che lo si possa risolvere con un emendamento al decreto fiscale. Chiedo a quest'Assemblea di porre attenzione a quello che accadrà dopo che questo emendamento sarà stato chiedo alla Commissione industria di approfondire l'argomento, perché parliamo di decine di miliardi di euro, parliamo di decine di migliaia di lavoratori parliamo della più importante infrastruttura di questo Paese, ovvero quella digitale. Spero che qualcuno in questa Aula mi abbia ascoltato.

È una questione di tale centralità per la modernità del nostro Paese e per la sfida competitiva dell'Italia, anche nel quadro europeo, che noi siamo interessati a incoraggiare il tema, la scelta di riorganizzazione, la resa univoca della rete digitale dell'Italia per l'Europa. Ma è curiosa e non è all'altezza della sfida la modalità con la quale siamo arrivati a prendere questa iniziativa e ad assumere questa potenziale decisione. C'è da definire la *par condicio* di accesso all'infrastruttura e occorre fare in modo che il diritto alla concorrenza caratterizzi l'utilizzo dell'infrastruttura. Noi siamo convinti che l'infrastruttura digitale rappresenti il futuro della sfida, non solo in Italia. Questo significa competitività per le imprese, per i territori, il superamento anche delle distanze che fino ad oggi hanno messo in difficoltà le città e anche l'intrapresa di chi vuole creare ricchezza dal punto di vista dell'economia. Ma quello che non va bene è che il sito normativo del decreto-legge fiscale è diventato tutto e il contrario di tutto. Noi in Commissione abbiamo molto incoraggiato la riflessione su questo punto. Abbiamo detto di scegliere un sedime normativo dedicato per valutare l'impatto non solo sul piano economico, ma l'impatto normativo riguardante tutti i siti che vengono coinvolti da questa rivoluzione strategica e digitale. Per questa ragione ci siamo astenuti in Commissione, nella speranza che in Aula ci fosse un soprassalto di univocità di lettura. Ci asteniamo anche in questa sede e diamo valore alle parole venute dal Gruppo Forza Italia, attraverso il parlamentare che è intervenuto, e speriamo che Governo e Commissione competente si ritrovino.

in cui il Senato approvò la risoluzione che il Governo avrebbe dovuto portare a Bruxelles, per far inserire nell'agenda

Oggi è presente il sottosegretario Bitonci, che credo conosca bene la questione perché ovunque, in ogni trasmissione televisiva, i rappresentanti della Lega o indossano la maglietta «no alla Bolkeistein» o fanno altri tipi di attività o prendono posizione. Su questo siamo d'accordo. Aspettiamo ancora

noi vogliamo sapere dal Governo quando volete sedervi al tavolo per risolvere la questione. Noi abbiamo già volte la disponibilità e ancora non abbiamo avuto l'opportunità di discutere con voi. Noi ci siamo. Credo che siamo arrivati alla fine della pazienza; non tanto noi come Gruppo parlamentare di Forza Italia, ma le imprese che vedono arrivare il 2020 e vedono portarsi via sessant'anni di lavoro, di storia e di esperienza familiare.

Lo ritiriamo perché ci riteniamo soddisfatti dell'accoglimento da parte del Governo in Commissione di un ordine del giorno che racchiude diverse problematiche che abbiamo sottoposto in questo provvedimento. Partiamo dalla problematica più rilevante, che ingloba tutte le altre che descrivo in ordine, relativa alle concessioni demaniali marittime; si tratta di una materia che attraversa, come diciamo ormai ogni giorni e come ha detto il collega di Forza Italia prima, un periodo di profonda incertezza per tutti i concessionari demaniali e per gli imprenditori del settore a causa di frettolosi interventi normativi imputabili ai passati Governi, che hanno abrogato alcuni principi di diritto senza procedere, in via preventiva o parallela, a introdurre le necessarie disposizioni normative sostitutive o correttive. Mi riferisco all'abrogazione del cosiddetto diritto di insistenza - precedentemente consacrato dall'articolo 37 del codice della navigazione navigazione - intervenuta nel 2010 per scongiurare ipotetiche posizioni di contrasto della normativa nazionale valevole nella materia della cosiddetta direttiva Bolkestein. Tutto ciò ha generato una situazione di profonda incertezza negli imprenditori balneari, che rappresentano oggi una fetta importantissima e considerevole dell'economia turistica nazionale. Si consideri che attualmente sono presenti 30.000 imprese circa che operano nel settore turistico-ricreativo-balneare turistico-ricreativo-balneare con tutte le conseguenze in termini numerici sull'economia dei singoli territori, sui livelli occupazionali garantiti, sugli indotti della filiera locale di prodotti di prodotti agroalimentari e sulla promozione del territorio attraverso la canalizzazione del turismo balneare verso altri interessi turistici di carattere culturale, enogastronomico e artigianale nel nostro Paese. A fronte di tale importante e comprovata rilevanza turistica ed economica, si inserisce anche la situazione più grave dell'incertezza normativa in merito alla durata dei titoli concessori, che ha spinto gli imprenditori balneari a stoppare qualsiasi iniziativa finalizzata a investire sulle proprie aziende. Negli ultimi anni le fiere di settore si sono ridotte a incontri e seminari con piccoli *stand* sempre minori e sempre più vuoti. È una materia che meritava e merita la giusta attenzione e di cui siamo convinti il Governo, tramite il sottosegretario Bitonci e il il nostro Ministro all'agricoltura e al turismo, si sta occupando. Presidente, come se non bastasse, negli ultimi periodi alcuni territori del nostro Paese sono stati colpiti da eventi climatici e atmosferici catastrofici, con danni ingenti al territorio e ai beni personali e delle imprese stesse. altrettanta importanza e attualità è la problematica che abbiamo inserito all'interno dell'ordine del giorno sulla materia balneare. Mi riferisco al mantenimento, per l'intero anno e non solo per la stagione estiva, di tutti quei manufatti funzionali alle attività turistiche e ricreative balneari ubicati su area demaniale, ovvero su proprietà privata. Permane su tutto il territorio nazionale l'impossibilità per la gran parte dei manufatti funzionali alle attività

assentiti con titoli stagionali. Tale situazione ha dato vita a un corposissimo contenzioso che ha visto nella gran parte dei casi vittoriosi gli imprenditori balneari, con conseguente danno alle casse dell'erario sul piano delle spese processuali. In alcune Regioni (come, per esempio, la Puglia) la stagionalità dei manufatti viene sistematicamente sancita anche laddove sussiste una legge regionale - mi riferisco alla legge regionale n. 17 del 2015 - che prevede il diritto al mantenimento annuale. La situazione ormai è all'assurdo e porta dei connotati particolarmente gravi e rilevanti. I concessionari, pertanto, si trovano nella condizione di dover promuovere lunghe azioni giudiziarie e di dover rimuovere le strutture al termine di ogni stagione,

anche in considerazione delle tempistiche necessarie per smontare la struttura e poi rimontarla dopo pochi mesi. Un ulteriore danno nel settore turistico che determina la situazione sopra evidenziata è rappresentato dall'impossibilità di poter garantire durante tutto l'anno l'apertura degli stabilimenti balneari, anche nell'ottica di una destagionalizzazione reale e concreta del turismo balneare, che i flussi turistici, soprattutto quelli stranieri, sono presenti nel nostro territorio nazionale durante tutto l'anno e non solo d'estate e risentono concretamente di una stagionalità della per questo motivo sarebbe opportuno e necessario un intervento normativo che autorizzi i titolari delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative che utilizzino manufatti amovibili a mantenere installati i predetti manufatti per tutto l'anno

Signor Presidente, chiedo scusa all'Assemblea se il mio intervento sarà di natura strettamente tecnica ma è mio desiderio che rimanga agli atti. Come sapete, stiamo per approvare un emendamento il cui fine è porre rimedio a un problema gravissimo che è stato determinato all'esito della sentenza della Corte di cassazione n. 18135 del 2015. In estrema sintesi, la sentenza ha stabilito che la vendita di taluni beni in regime di edilizia convenzionata, in violazione dei limiti di prezzo, determina la nullità parziale del contratto per la quota esuberante rispetto al prezzo cosiddetto calmierato. Segnalo che la Corte di cassazione ha ritenuto di concludere *tout court* per la nullità, senza svolgere un'indagine sull'interesse protetto dalla norma. È noto che la nullità assoluta del nostro ordinamento entra in gioco nel caso in cui l'interesse protetto sia sovraindividuale e indisponibile. Che l'interesse in questione sia disponibile è confermato dal fatto che la norma già in vigore consente di eliminare tali vincoli tramite l'affrancazione, quindi trattasi non di un interesse indisponibile, ma di un interesse assegnato alla disponibilità dei privati, ancorché di rango pubblicistico. Dunque, la sanzione della nullità appare ultronea rispetto alla *ratio* della norma. Sul punto dunque interviene quella che si definisce un'interpretazione autentica del legislatore. Ricordiamo che la norma originale non indica espressamente la nullità, che è frutto di un combinato disposto. Qui l'interpretazione autentica del legislatore indica nella parziale inefficacia del contratto, limitatamente alla quota esuberante di prezzo, la conseguenza della violazione della norma stessa, con delle conseguenze importanti dal punto di vista sistematico, giacché evidentemente la patologia dell'atto può essere sanata dal venditore nel caso in cui questi provveda ad attivare il procedimento, ancorché *ex

accennato qualche attimo fa all'emendamento 25.0.18, che era stato ritirato. O sbaglio? PRESIDENTE. Ci sono una serie di emendamenti aggiuntivi all'articolo 25.

su cosa intervenuti. Posso chiederle di cosa stiamo parlando in questo momento?

che riguarda la possibilità di concedere degli incentivi all'acquisto di veicoli ibridi ed elettrici. Riteniamo che la sensibilità ambientale dovrebbe, almeno a quanto si proclama, essere trasversale a questa quindi mi appello davvero brevemente a tutto il Senato affinché ci ripensi e dia voto favorevole per favorire l'ambiente e per favorire anche un settore economico importante come quello dell'*automotive*.

nei presidi socio-sanitari, socioassistenziali e socioeducativi di poter lavorare anche nei presidi sociosanitari in cui già lavorano da molti anni

favorire il miglioramento dell'offerta dei servizi sociosanitari, socioeducativi e socioassistenziali e, dall'altro, di non estromettere del personale, e sto parlando di circa 150.000 operatori che già lavorano,

Signor Presidente, vorrei sottolineare l'importanza di questo emendamento, che riguarda la questione della direttiva Bolkestein applicata agli stabilimenti balneari. balneari. Posso comprendere che, anche per un sano esercizio di realismo, la maggioranza abbia appena respinto una serie di emendamenti che tendevano a risolvere il problema, ma che avevano una onerosità dal punto di vista del bilancio, tant'è che la 5a Commissione aveva Commissione. In questo caso, invece, siamo in presenza di un emendamento che va incontro ad una posizione che credo sia largamente condivisa all'interno del Parlamento. Si di un emendamento che prende spunto da una recente sentenza del Consiglio di Stato che ha chiarito che, proprio sulla base della direttiva Bolkestein,

tuteli gli stabilimenti o comunque offra anche al Governo uno strumento in più per tutelare gli stabilimenti. Il ministro Centinaio è impegnato su questo fronte e sappiamo che ha aperto un tavolo di confronto con le categorie che attualmente sta lavorando al Ministero. Noi crediamo che approvare questo emendamento aiuti il ministro Centinaio e il Governo: se davvero si vuole risolvere il tema della Bolkestein e tutelare Grazie, spunto da una sentenza del Consiglio di Stato nonché esattamente dalle deroghe previste dalla direttiva, quindi in perfetta coerenza con le sentenze dello Stato e con le direttive europee, inserisce uno di rafforzamento e di tutela verso l'azione del Governo. Chiedo al relatore e alla maggioranza di riflettere sull'emendamento 25.0.37 e di volerlo accogliere, perché faremmo tutti insieme un passo avanti positivo verso la soluzione di un problema che credo stia cuore non solo a Fratelli d'Italia, ma a una larga maggioranza o almeno a una qualificata maggioranza di questa Camera.

del territorio e in questo Parlamento e da parte del Governo. È un emendamento che finalmente dà la possibilità a dei lavoratori che ad oggi erano stati

ai lavoratori che, purtroppo, sono stati estromessi dal ciclo produttivo a causa di aziende che, vista la crisi, hanno cessato. Difatti, ricordiamo il ripristino, da parte di questo Governo, della cassa integrazione

desidero sottolineare l'importanza di questo emendamento, perché finalmente si torna all'incompatibilità tra una figura istituzionale e il commissario *ad acta* in sanità, quindi non vi sarà più un doppio incarico e il Governatore di una Regione non sarà più il commissario *ad acta* per *(Applausi dal Gruppo M5S)*. L'esperienza degli ultimi anni è evidente a tutti, ogni settimana leggiamo sui giornali cosa succede in queste Regioni: faccio l'esempio della Campania, con De Luca, faccio l'esempio della Campania, con De Luca, e della Regione Lazio, dove lo stesso Zingaretti da mesi informa tutti che stiamo per uscire dal piano di rientro, ma ancora non siamo usciti. Quindi, mai più il doppio ruolo.

nonché specifica esperienza nell'ambito di gestione della sanità, con particolare riguardo alla legalità e all'anticorruzione. quindi che capirete l'importanza di questo emendamento per migliorare la sanità nelle Regioni in cui i tagli l'hanno praticamente uccisa.

anche dei grandi diritti che hanno accompagnato la popolazione italiana, le fasce medio-basse: il diritto al lavoro, all'istruzione e il diritto alla salute appena richiamato dal collega Sileri.

che questo Stato ha degnamente rappresentato nel corso degli anni, con i suoi successivi Governi. Come diceva poc'anzi, in un precedente intervento, il collega Grassi, che ha espresso tecnicamente un

dove c'è stata, purtroppo, una dimenticanza da parte dello Stato. Queste famiglie sono state abbandonate...

anche al Partito Democratico, che ha presentato un emendamento (poi ritirato e ripresentato come ordine del giorno) che ricalca esattamente il testo del nostro emendamento, di condividerlo, anche per dare un po' il segno a quei cittadini, che vorrebbero non sentirsi più abbandonati da tutti noi, che siamo in grado di intervenire immediatamente. Voglio contestualmente ringraziare, proprio perché è stata un'azione estremamente condivisa, a partire dall'interlocuzione iniziale con i cittadini e con i comitati che li rappresentavano, Scusi, signor Presidente.

qualunque persona intervenga, non ha mai nessun problema di inopportunità, diversamente da chi, precedentemente, è intervenuto in quest'Aula.

questo ormai è diventato un decreto *omnibus* e su questo vorrei porre la prima questione, in quanto è la prima ragione del nostro voto contrario. Ormai è diventata una prassi. Questa, dicevo, è la prima ragione del nostro voto contrario. Ormai la forma che ha assunto il modo di rapportarsi del Governo con il Parlamento è segnata da questa particolarità. Oddio, non è che sia una novità, è una sottolineatura, però.

le Commissioni che non hanno il tempo per approfondire e che vengono convocate e sconvocate. Poi c'è la rincorsa tra MoVimento 5 Stelle e Lega a marcarsi su questo o quel posizionamento, forse elettorale, ma questo sequestra il lavoro delle Commissioni e del Parlamento. le parole pronunciate dal Presidente del Consiglio e pronunciate da tanti rappresentanti della maggioranza sul rispetto del Parlamento e delle prerogative del Parlamento sono parole assolutamente al vento. In ogni caso, affrontare questioni rilevantissime, come ad esempio quella della rete, di cui si è parlato prima, in questo modo è un gravissimo danno non solo al confronto tra opposizione e maggioranza, ma anche all'approfondimento del lavoro. Da questo punto di vista, vorrei invitare con tranquillità il Parlamento, ma soprattutto il Governo e la maggioranza, a fare una riflessione. Io non ho mai detto che questa maggioranza e questo Governo sono fatti di persone incompetenti. Tuttavia, la scienza in tasca non l'avete neanche voi e sarebbe utilissimo un confronto di merito, nelle sedi istituzionali, tra la maggioranza e l'opposizione. Forse converrebbe anche a voi, per evitare errori che già in altri provvedimenti avete commesso. il relatore, e non solo il relatore, ha detto che si è realizzato, con questo provvedimento, un nuovo rapporto tra fisco e cittadini: no, non è vero, non è assolutamente vero. Questo Governo percorre la più classica strada percorsa in tanti anni da tanti diversi Governi dirò la parola che tanto dà fastidio a molti colleghi della maggioranza: la strada del condono. rappresentanti del MoVimento 5 Stelle hanno detto che non è un condono. Esatto, non è un condono: sono più condoni, più condoni, che peraltro non risolvono nemmeno il problema in nome del quale parlate di pace fiscale, perché non affrontate

vorrei dire con chiarezza, a proposito di Governo del cambiamento: voi fate norme condonistiche di sanatoria, puntualmente identificando categorie e vostri potenziali elettori. Non siete nel Governo del cambiamento, siete nel solco classico che ha governato - ahimè questo Paese lungo questi quarant'anni e su questa strada non farete nessun passo in avanti. Ma la cosa più grave

due piccole imprese su tre pagheranno più tasse (è chiaro? Pagheranno più tasse!). che nemmeno dal punto di vista delle entrate ottenete un risultato positivo. Da questo punto di vista, è sostanzialmente un capolavoro. ciò che davvero va sottolineato è che il vostro discorso ha disperso - lo dico anche ai ai colleghi e alle colleghe del MoVimento 5 Stelle - la lotta all'evasione fiscale. Ora, noi siamo un Paese singolare. Quando si fanno i convegni e i comizi, la lotta all'evasione fiscale è al primo posto cosa succede quando si va al merito e si fanno queste discussioni? Badate bene, io non sono tra quelli che pensano che i lavoratori autonomi siano evasori, ma parliamoci chiaro: se la Banca d'Italia parla di 103, 108, 120 miliardi di mancate entrate per l'erario, chi è che evade? C'è qualcuno che evade? C'è un problema da porsi? Il vero discorso serio da fare sarebbe: si pagano troppe tasse! Sì, troppe tasse per chi le paga, per chi ha la trattenuta alla fonte e per i cittadini onesti che nelle imprese - e ce ne sono tanti - pagano tutte le tasse. Il discorso che voi state facendo al Paese è un discorso che non è in grado di elevare quel senso civico di fedeltà fiscale e il messaggio che voi mandate è un messaggio che incita. e alla rottamazione-*bis*: perché devo pagare, se so che poi arriva un altro provvedimento che mi darà condizioni migliori di quelle di prima?

Sono certo, al di là del racconto, al di là della demagogia, al di là del fatto che in questo Paese nessuno evade, al netto di quei 108 miliardi di evasione, che alla fine state procurando un danno e lo dico a chi, giustamente, parla della necessità di rafforzare la funzione pubblica e la funzione dello Stato. È difficile così parlare di giustizia fiscale e, alla fine, tutti i discorsi stanno a zero. Vi sono poi alcune proposte di emendamenti che noi abbiamo fatto, regolarmente respinte. Presidente, si parla di autonomia speciale per le Regioni, ma avete respinto tutti gli emendamenti che tutelavano l'autonomia delle Regioni e dei Comuni.

Che fine fa l'autonomia, se non lasciate nemmeno lo spazio a un Comune di decidere se vuole rottamare o meno le cartelle sui propri tributi?

fondamentale che sorregge la vostra campagna sull'immigrazione. Voi dite: aiutiamoli a casa propria. In verità, non poteva mancare (perché ormai va in automatico, è nel programma di iscrizione di tutti i provvedimenti) una norma contro gli immigrati. Fissate una tassa sulle rimesse. Aiutiamoli a casa propria, ma solo un po'. Queste persone sono immigrati regolari, che quando fanno il trasferimento delle risorse (le rimesse) pagano già l'8 pagano le tasse, contributi per pensioni che non vedranno mai e che non riceveranno mai indietro; e voi, che li volete aiutare a casa propria,

Signor Presidente, dopo i numerosi interventi che ho potuto fare in quest'Aula in discussione generale e in sede di illustrazione dei singoli emendamenti, nei quali mi sono anche accalorato per l'importanza dei temi che abbiamo trattato, mi sembra corretto e doveroso esordire in questa dichiarazione di voto sottolineando, in particolare, il clima costruttivo che comunque ho potuto riscontrare nella Commissione finanze,

il decreto-legge fiscale e, più in generale, la manovra di bilancio del vostro Governo devono essere letti nella contrapposizione tra due termini che, nel pensiero comune e spesso in tanti politici come noi, vengono considerati come concetti equivalenti: quello di sovranismo e quello di populismo. In effetti, però, sono due concetti che identificano realtà ben diverse. Noi siamo fieramente sovranisti; non siamo e non saremo mai populisti. Purtroppo la lettura che io do di questo decreto-legge e, più in generale, almeno per ora, per quello che mi è noto, dell'intera manovra di bilancio,

ma guardano piuttosto alla pancia della persona, al bisogno immediato, attuale del cittadino. Insomma, è un po' la distinzione che c'è oggi tra il politico e la politica, tra la politica che grida necessità di guardare al futuro, di avere una strategia e il politico che, invece, guarda solo al contingente, ad andare sui giornali, a rispondere ai bisogni immediati della persona. Ecco, su questa contrapposizione va letta anche questa manovra di bilancio.

e che chiedono una visione strategica a coloro che sono demandati a fare leggi e atti di Governo. Fratelli d'Italia ha cercato, nell'attività in Commissione e in quest'Assemblea, di darsi un'impronta costruttiva. Non abbiamo fatto ostruzionismo; non abbiamo criticato solo per criticare, ma abbiamo cercato di dare un risvolto di crescita a questo decreto-legge. Abbiamo cercato di far sì che quei 10 miliardi destinati all'assistenzialismo potessero, almeno in parte, essere rivolti alla crescita, cioè essere destinati alle nostre imprese, alle piccole e medie imprese italiane, al lavoro, al cuneo fiscale e ai nostri lavoratori. Abbiamo, cioè, cercato che quei soldi, destinati all'assistenzialismo,

obiettivi e stimoli, dando lavoro, facendo lavorare i nostri giovani, dando loro delle opportunità che saremo in grado di avere una Patria e un'Italia migliore. Su questi fronti ci siamo impegnati impegnati e abbiamo ottenuto qualche piccola soddisfazione con l'approvazione di tre emendamenti in sede di Commissione, con l'ottenimento del *placet* del Governo. Saremo attenti a verificare se quest'ultimo prenderà atto dei nostri sei ordini del giorno, che spaziano su vari temi, dalle quote latte (che interessano i nostri agricoltori), fino ad altri aspetti, come quello del credito cooperativo. cooperativo. Ne ho parlato a lungo in questi giorni, ma permettetemi ancora una sottolineatura: è stato abbandonato a se stesso e, quindi, l'unico gruppo bancario nazionale, quello delle banche del Credito Cooperativo e Casse Rurali, è oggi lasciato in balia della finanza internazionale.

si è determinata una piccola pacificazione. Ovviamente prendiamo atto e apprezziamo che si siano date delle risposte alle cartelle esattoriali, a qualche processo verbale che si potrà definire e che si sarebbe potuto definire meglio e che, invece, non si è voluto fare. Accettiamo e condividiamo qualche passaggio, però ricordiamo, innanzitutto, che una pacificazione fiscale ha un senso nel momento in cui si accompagna a una riforma

una forma di condono ai contribuenti per uscire dal contenzioso. Così non è stato. È stata solamente una piccola pacificazione che sarà inadeguata a fare cassa perché, come ho già anticipato, non porterà ciò che ci si aspetta.

povero contribuente vessato dalle cartelle - ripeto: ben venga - nascondendo magari dietro a questo delle misure che hanno reso il sistema tributario italiano ancora di più il Grande Fratello fiscale, uno Stato di polizia fiscale. Ricordiamoci che da domani, grazie al decreto-legge in esame, la Guardia di finanza potrà guardare nei conti correnti di ciascuno di noi senza nemmeno aver avuto preventivamente l'assenso della procura della Repubblica.

onesti e coerenti con i propri ideali, affinché sappiano rivedere qualche posizione e dare una risposta davvero coerente con le necessità del Paese, dei cittadini e del mondo delle imprese.

il decreto fiscale - è stata l'ennesima occasione per demolire il senso dello Stato, già fortemente incrinato dalle vostre promesse. Poteva essere il momento per parlare seriamente di molti dei temi che avete aggiunto dopo, in Commissione e a volte in Aula. Tuttavia, il peso di questo condono, che è il tratto di fondo della proposta che avete presentato, resta determinante rispetto agli altri temi e, per questo, inaccettabile. Nei testi di scienza delle finanze si legge che l'evasione fiscale indica tutti quei metodi volti a ridurre o eliminare il prelievo fiscale da parte dello Stato sul cittadino contribuente, attraverso la violazione di norme fiscali da parte di quest'ultimo. Costituisce di fatto - continuano i testi di scienza delle finanze - un fenomeno deleterio e contribuisce a far perdere allo Stato una parte non trascurabile delle entrate, creando debito pubblico e mancati interventi per la crescita economica. Questa è l'evasione fiscale. Sotto la voce pace fiscale, di cui vi siete riempiti molto spesso la bocca, non esiste alcuna spiegazione. È solo una vostra invenzione lessicale, nulla di più. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Chi evade rompe il vincolo di solidarietà con la comunità e fa pagare agli altri il prezzo del proprio illecito arricchimento. E chi sono questi altri che pagano? Sono i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, i pensionati, i lavoratori autonomi e gli imprenditori onesti. Sono questi che pagano, prima e dopo il condono. È nella tassazione che si manifesta quel felice connubio tra lo Stato e il contribuente, attraverso un patto: lo Stato fornisce servizi e il contribuente paga parte di questi servizi e partecipa (ovviamente servizi che siano di qualità). il Governo, anziché contrastare il fenomeno che riduce i servizi e aumenta il debito pubblico che cosa fa? Con un condono favorisce coloro che non partecipano a questo patto. Esattamente il contrario di quello che dovrebbe fare. Sono noti quelli che pagheranno, li abbiamo elencati. Ma chi sono i contribuenti interessati dal decreto-legge? Chi sono questi signori che potranno usufruire del condono fiscale di cui parlate? Sono coloro verso i quali è stato elevato un verbale di constatazione o hanno già ricevuto un avviso di accertamento o hanno una lite pendente fino in Cassazione con il fisco. Non avete dimenticato nessun passaggio amministrativo, pur di premiare i furbi. Non ci sono altre ipotesi nel campo tributario per premiare coloro che hanno evaso. I processi verbali di constatazione, com'è noto, sono quelli che concludono l'attività fiscale e nel quale sono contenute le sanzioni e i vari tributi da pagare. Ebbene, con un colpo di spugna, voi date la possibilità a coloro che sono stati beccati dal fisco, presi con le mani nella marmellata, di condonare tutto, di sanare quello che hanno evaso. A questo proposito, mi permetto una digressione. Colgo l'occasione offerta dalla quotidianità e ringrazio la famiglia Di Maio per aver offerto questa possibilità. Per l'arricchimento da lavoro nero - e così faccio un riferimento a colui che stamattina impropriamente l'ha detto nei nostri confronti - alla società di famiglia seguirà certamente l'accertamento fiscale e tributario certamente si concluderà con un rilievo positivo; almeno questi: dichiarazione infedele, irregolarità formali, mancati versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. Ebbene, se queste violazioni fossero state scoperte un anno fa, il signor Di Maio avrebbe potuto usare il vostro condono per sanare tutte le violazioni che ha commesso. Guardate il segno del destino. Che caso! Scoprire che la famiglia del Vice *Premier* del nostro Paese poteva, se fosse stata scoperta un anno fa, usufruire del condono che che oggi voterete in quest'Aula. È un vero e proprio premio per chi ha evaso. Questo è il decreto-legge. Il vostro regalo difficilmente si spiega con la necessità di fare cassa. Non credo. Si spiega dal punto di vista culturale: avete manifestato una visione malata dello Stato che umilia gli onesti e chi rispetta le regole pur di premiare i più furbi. Ma questo contribuente, spesso è stato detto in Commissione, è un presunto innocente o è un colpevole evasore? Con il verbale di constatazione è un presunto innocente può ricorrere fino al terzo grado di giudizio, ma nel momento in cui accetta il vostro condono e presenta la dichiarazione di partecipazione, diventa colpevole di evasione fiscale. Lo dico a chi ci accusava in Commissione di giustizialismo dal punto di vista fiscale. con verbale di constatazione diventa, per voi, evasore fiscale perché accetta di condonare e se questo signore ha nascosto altri redditi che l'amministrazione finanziaria non è stata in grado di accertare con il processo verbale di constatazione, nessun altro potrà andare a vedere i suoi conti per gli anni che condonerà, la farà franca su tutti i redditi che ha evaso, non solo quelli per i quali è stato verbalizzato. Andiamo avanti. Altro che favorire - mi viene in mente un intervento di ieri - la crescita trovando le risorse: voi le regalate, le risorse, a chi ha evaso, peraltro.

È stato detto che l'evasione di necessità è di colui che presenta la dichiarazione e poi non è in grado di versare i contributi e le imposte che avrebbe dovuto pagare. E questo provvedimento l'affronta? Assolutamente no. Avete usato una narrazione che persuade. Eravamo anche disponibili ad affrontarla, ma nel decreto-legge non c'è assolutamente nessuna misura che si dimostri a favore dell'evasione cosiddetta di necessità. Avete utilizzato questa narrazione retoricamente per premiare coloro che invece sono più furbi e l'hanno fatta franca. Non è un'evasione di necessità quella di chi viene verbalizzato perché nasconde i suoi redditi e non perché non riesce a pagare le imposte. Tra un condono e l'altro, avete inserito anche una tassa, la tassa di 200 euro per gli errori formali, con un'assurdità: tutti gli economisti sanno che le sanzioni per le irregolarità formali sono singole, per voi una, 10, 1.000 irregolarità formali saranno sanate con 200 euro, nulla di più. È così vero che è una tassa, che la somma di tutte le irregolarità sostanziali sanate con gli altri articoli ammonta a circa 600 milioni di euro, mentre solo con questo articolo le irregolarità formali garantiscono 1,3 miliardi in due anni. Lo sappiamo come funziona in Italia: anche l'onesto, per non avere problemi, sosterrà la spesa di 200 euro (100 l'anno prossimo e 100 nel 2020) per sanare la sua posizione. E che dire dello stralcio dei debiti fino a 1.000 euro? Tanta attenzione verso gli evasori e nessuna considerazione per gli enti locali che perderanno risorse senza alcun ristoro. Questo è davvero stucchevole: da una parte i Comuni che perderanno soldi e dall'altra gli evasori che la fanno franca. A corollario dello scempio fiscale del condono, che è diseducativo e depressivo per l'erario, ricordo la chicca della sanatoria per le sigarette elettroniche (anziché seguire una sentenza della Corte costituzionale, sanate tasse per 177 milioni di euro) avete cancellato, appunto, tutte le tasse dovute, nonché la pervicace volontà di destrutturare e depotenziare una infrastruttura strategica del nostro Paese qual è quella fiscale della fatturazione obbligatoria.

avete abbandonato la strada della lotta all'evasione e all'elusione, avete calpestato lo statuto del contribuente che tanti risultati positivi ha garantito in questi anni e avete iniettato il *virus* della malafede e del condono, che premia i furbi e rende alcuni contribuenti più uguali degli altri. Questo è sbagliato in uno Stato di diritto. Il condono è un tratto distintivo di questo Governo. Pensate che su quattro decreti-legge, quelli più importanti che abbiamo affrontato anche in quest'Aula, due si riferiscono a un condono (edilizio per Ischia e fiscale come quello che stiamo affrontando Credo sia un *record* negativo mai visto nella storia della nostra Repubblica che il 50 per cento dei vostri provvedimenti affrontati finora sia riferito a condoni (fiscale e edilizio): una vergogna. Oggi siamo convinti, in ragione di queste considerazioni che ho espresso, che avete reso lo Stato ancora più debole e continuerete, da quello che si capisce e da quello che sentiamo, su questa strada.

Signor Presidente, gentili colleghi, ho accettato con gratitudine l'incarico del Capogruppo di esprimere la dichiarazione di voto del mio Gruppo sul decreto-legge fiscale: un provvedimento che ho accompagnato nel suo percorso in 6a Commissione al Senato. Ringrazio i colleghi che hanno generalmente espresso un apprezzamento per il modo con cui abbiamo cercato in quella sede di dare alle nostre opposizioni la possibilità di esprimere il loro contributo. Voglio anche esprimere un ringraziamento non di circostanza agli Uffici, che ci hanno aiutato nel compito complesso di affrontare un provvedimento che, per le sue sfaccettature, necessitava di un supporto consistente, anche sotto il profilo tecnico. Quando mi sono affacciato al mondo della politica, l'ho fatto portando con me le parole di un amico, Giorgio La Malfa, che mi aveva detto che questa esperienza mi avrebbe arricchito culturalmente. Credo che volesse dirmi che avrei visto tante cose strane. In effetti, questo, in qualche modo, sta succedendo. Una l'ho vista oggi, quando mi sono sentito rimproverare la mancanza di autonomia valutativa

ad apprendere è piuttosto impegnativo, per dare prova di autonomia, se non valutativa quantomeno discorsiva, non ho con me un foglio (perché non ho avuto il tempo di scriverlo, essendo tante le questioni da affrontare). Voglio quindi soffermarmi, con con spontaneità, sincerità e con lo spirito di confronto che ha caratterizzato un po' tutta la genesi del provvedimento in Commissione, su tre punti su tre punti che mi sembrano essenziali, sui quali mi piacerebbe veramente che, posatasi la polvere e attenuatisi i toni, che sono necessariamente accesi in Assemblea, si possa riflettere con calma. Un punto è il contesto; un altro è il metodo e un terzo punto sono i contenuti. Il contesto nel quale questo decreto-legge nasce è stato evocato dalla collega Conzatti, relatrice di minoranza, facendo, però, riferimento alle informazioni giornalistiche degli ultimi giorni e delle ultime settimane, che dipingono un'Italia completamente allo sbando; un Paese sull'orlo della bancarotta per colpa di noi, i barbari. Vi proporrei, tuttavia, un esercizio diverso. Per apprezzare il tipo di operazione che è stata fatta con questo decreto-legge, vi proporrei di allargare un po' lo *zoom* e magari di non rifarci alle fonti della stampa, che necessariamente esprime un ampio ventaglio di opinioni, ma, come sapete, citando - visto che qualche giorno fa abbiamo commemorato un grande classico del nostro cinema - un classico del cinema statunitense, l'ispettore Callaghan, le opinioni ognuno ha le sue. Io vorrei piuttosto soffermarmi sui dati - guardiamo cosa ci dicono - secondo cui ci vorranno ancora cinque anni perché il livello del reddito in Italia ritorni a essere quello pre-crisi. Questa frase ve l'ho già detta in altre circostanze, quindi rischia di diventare un ritornello un po' stantio. Per arricchirla di icasticità, mi sono permesso di mettere il grafico sul mio *blog* così chi vuole può andare a vederlo, sta lì. Ci vorranno altri cinque anni, e questo non significa che fra cinque anni la crisi sarà finita: significa che fra cinque anni avremo anni di ritardo sulla nostra storia. Significa che, nella storia del prodotto interno lordo di questo Paese, la crisi appena terminata ha aperto una cicatrice che si vedrà per i prossimi secoli, se qualcuno fra secoli avrà voglia di registrare ancora il PIL come oggi lo concepiamo. L'evento nel contesto del quale ci muoviamo muoviamo in termini economici ha la dimensione di un evento bellico. Questo per dire che, quando sento porre questioni pregiudiziali rispetto all'urgenza d'intervenire in campo fiscale, non posso resistere alla tentazione di considerare queste eccezioni come strumentali o come derivanti da un non completo apprezzamento della tragicità della situazione nella quale siamo, della drammaticità della situazione del nostro Paese. Questo per il contesto. ricordare che altri Paesi, i quali a differenza di noi non hanno ritenuto di fare i primi della classe obbedendo a tutte le regole dettate dai loro concorrenti, hanno già raggiunto - e anche questo lo trovate oggi sul mio *blog* - il sentiero di crescita di lungo periodo. Fra il sentiero di crescita pre-crisi e quello sul quale siamo adesso c'è un *gap* di 400 miliardi di euro, che non so se riusciremo mai a recuperare. Teniamo conto di questo quando parliamo di un atteggiamento condonistico.

in Commissione finanze il senatore D'Alfonso, del quale anche in questa sede abbiamo potuto apprezzare l'eloquenza, che comunque è sempre pregna di contenuti e ci permette di approfondire l'analisi.

siamo dovuti intervenire anche perché c'è una storia di provvedimenti di struttura presi in un sedime normativo inadeguato. Noi abbiamo cercato di rimediare ad alcune criticità emergenti da riforme del credito fatte per decreto-legge, senza una necessaria adeguata attività istruttoria ed eccependo un'urgenza che in quei casi invece non c'era. Infatti, se prendiamo ad esempio il comparto del credito cooperativo e andiamo a vedere cosa ne dicono le relazioni della Banca d'Italia, da nessuna parte emerge una necessità ed un'urgenza d'intervento complessivo in quel comparto. E quando poi si interviene

che una riforma, quella delle banche popolari, adesso è *sub iudice* alla Corte di giustizia dell'Unione europea per il semplice motivo che qualcuno ha riflettuto sul fatto che neanche i regolamenti europei sono così draconiani da prevedere che chi affida i propri risparmi a un istituito non venga rimborsato mai, che è l'interpretazione data qui in Italia di una regola europea. Ci sarebbe quindi da aprire anche un dibattito sul metodo, su questa nostra velleità di applicare sempre ciò che viene dall'estero in modo estremamente penalizzante per noi stessi. Fino a che noi non apriremo un dibattito

dai nostri concittadini, dai lavoratori italiani, più come una volontà di aggressione nei loro riguardi, che come una volontà di aderire a un progetto di ordine superiore. *(Applausi

A mia figlia a scuola hanno insegnato che gli articoli più importanti della prima parte della Costituzione sono il decimo e l'undicesimo, perché sono quelli che ci hanno consentito di entrare in Europa. Questo le è stato detto, poverina. Io non l'ho contestato, perché per carità! Non sia mai per me entrare nei percorsi didattici degli insegnanti. Però anche l'articolo 3 non è male. Lo vogliamo leggere insieme? «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». *(Applausi dai L'austerità, intaccando questi inderogabili doveri di solidarietà, ha messo, quella sì, a rischio il patto sociale del Paese. E che al termine di un periodo in cui abbiamo visto aumentare i poveri si ricorra a interventi di rottamazione che, a differenza dei precedenti, sono più accessibili (perché prevedono una maggiore dilazione delle rateizzazioni), quindi offrono un effettivo ristoro, non mi sembra che ci possa essere imputato come una grave violazione del patto sociale o come un sociale o come un aggiramento dei doveri che il contribuente ha nei riguardi dello Stato. Dobbiamo capire a che punto siamo: siamo in una situazione di estrema, tragica recessione, della quale - ahimè - non riusciamo a vedere effettivamente la fine. E proprio per questo motivo riteniamo - parlando di una cosa della quale qui oggi non si tratta - che l'impianto espansivo della legge di bilancio abbia una piena legittimità di essere e possa contribuire a risolvere il problema. È per questi motivi che dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito

il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame è una prima fase della manovra; potrebbe essere un collegato anticipato della manovra per il triennio 2019-2021. Il Governo con esso precorre la propria politica di bilancio facendo entrare in vigore da subito la propria idea di fisco. E anche la legge di conversione, probabilmente - uso il termine «probabilmente» perché ci sono voci anche di accorpamento rispetto alla manovra - anticiperà di quasi un mese la legge di bilancio. Ma i numeri di questo decreto-legge, anche dopo le modifiche introdotte, sono una cosa secondaria rispetto alla filosofia cosa secondaria rispetto alla filosofia che sottende, che non condividiamo, perché è solo la continuazione di quella dei Governi precedenti. Non possiamo accettare da parte nostra che la *ratio* possa essere quella che non si possa intervenire per semplificare e ridurre le incombenze, quali ad esempio la fattura elettronica, perché fanno parte di una misura che genera gettito già previsto dalla legislazione vigente e che altrimenti verrebbe a mancare. Di fatto si dice: non è per sviluppare il Paese, non è per agevolare le imprese, non è per fare un bene, ma è solo per fare cassa. Questa è la logica che sottintende l'articolo 10 del decreto-legge, *(Applausi dal Gruppo Per noi deve essere il contrario: quella che deve essere la finalità in un decreto fiscale è agevolare l'impresa, naturalmente di fare gettito per lo Stato, ma il gettito per lo Stato è l'agevolazione dell'impresa; la vostra posizione, richiamando la fatturazione elettronica quale strumento per far cassa, sottintende l'idea che questo Esecutivo *sui generis* ha del mondo produttivo e l'importanza che attribuisce alle piccole e medie imprese nel processo di crescita praticamente nullo. Non a caso, vorrei ricordare che le organizzazioni della grande impresa, che non ha problemi sulla fatturazione elettronica, non hanno nemmeno preso parte al confronto sul provvedimento.

e che può liberare, date da centinaia di migliaia di piccole e medie imprese, da professionisti, da lavoratori autonomi. Era questo il meccanismo basilare. Si è persa l'occasione, in sostanza, nel primo vero provvedimento fiscale che questo Governo ha posto in di togliere ogni incombenza possibile affinché costoro potessero dedicarsi alla loro principale ragione di vita, che è proprio il lavoro. La fattura elettronica a costoro non semplifica la vita: ora è così.

la riforma fiscale, quindi la *flat tax*, poi la creazione della rete, quindi la possibilità di utilizzo delle strade, e naturalmente il passaggio successivo è la fattura elettronica. Colleghi, è come se avessimo imposto l'automobile a chi non ha ancora la strada per viaggiare e ha solo il sentiero per farci passare l'asino. Questa è la sostanza della fattura elettronica per alcuni di costoro. Purtroppo il provvedimento contiene anche una serie di disposizioni in continuità con una politica fiscale «rapace e vessatoria»: non è una mia definizione, ma presa a prestito dall'intervento di ieri del collega Lannutti. Per il nostro fisco «rapace e vessatorio» adesso si aggiunge la possibilità, da parte della Guardia di finanza, di accedere ai conti correnti, che è tipico di governi che non sono quelli delle democrazie, ma dei totalitarismi.

non è più adeguata al nostro tempo. Perfino la progressività va a colpire solo chi produce, le imprese di fascia piccola e media e i lavoratori dipendenti. Non colpisce la grande impresa, non colpisce i grandi capitali e non colpisce i ricchi. Dobbiamo renderci conto della realtà e

il programma del centrodestra presentava la *flat tax* per far crescere il Paese e spiace che sia stata praticamente abbandonata, se non per una quota minima Non a caso, i Paesi che al mondo crescono in misura maggiore hanno adottato la tassa piatta. Va ricordato, peraltro, che con questo provvedimento i nuovi regimi, già previsti per il 2019, vengono abrogati e modificati ed è una caratteristica di legiferare che certamente non piace. Credo non piaccia all'opposizione, ma non piace nemmeno alla maggioranza. L'intervento del collega Bagnai mi conforta e, anzi, esprimo al collega Bagnai,

Quindi staremo sempre dalla parte del lavoro ed essere dalla parte del lavoro vuol dire anche rimarcare come

Non c'è riduzione della pressione fiscale. È vero, siamo usciti da un lungo periodo di crisi e abbiamo una situazione di difficoltà di credito, ma questo tipo di misure non fanno che accentuarlo. Le persone più attive nel nostro tessuto sociale, coloro che ogni giorno si alzano per andare a lavorare da dipendenti, oppure aprono la bottega o lo studio, devono confrontarsi con una situazione di calo dei volumi

dovuto prevedere la semplificazione e comunque un'attenzione per coloro che onestamente hanno dichiarato le imposte e non riescono a pagarle. Era questa la pace fiscale. Apprezziamo che sia stato approvato l'ordine del giorno a prima firma del nostro presidente Bernini, che impegna il Governo a porre attenzione a queste situazioni, ma l'ordine il giorno, che secondo il detto non si nega a nessuno, non è un provvedimento efficace. Quindi ritengo che non dobbiamo nemmeno cadere nel ragionamento di colpire, sparando nel mucchio, basandoci sugli 871 miliardi

provvedimento si chiama "fiscale", ma di fiscale sono rimasti nove articoli e per il resto c'è di tutto. Rimarco l'intervento sulla banda larga, che avrebbe dovuto prevedere una discussione e spero che ci sia ancora discussione nella Commissione di merito.

Vorrei ricordare - visto che viene sempre ricordato anche nei dibattiti televisivi, anche dal presidente Conte, che ci sono 17 miliardi di euro investimenti - che ci sono 16,5 miliardi di euro di investimenti, ma ci sono 39,5 miliardi di euro in più di spesa corrente e 74 miliardi di euro di debito aggiuntivo. Questo è il risultato complessivo dell'azione,

ripartire dalle persone, ripartire dalla società, ridare una possibilità alle persone perbene, che sono inciampate: la sfida affascinante che il Governo ci lancia e che la maggioranza raccoglie. Ripartire dalle persone perbene. Del resto, a cosa serve la politica quando si deve curare soltanto della stabilità finanziaria, che è importante,

Anche con il decreto fiscale in esame ripartiamo dalle persone, dai cittadini e magari da quei piccoli contribuenti, da quelle piccole imprese che loro malgrado non sono riuscite a

In manovra abbiamo messo il reddito di cittadinanza, per dare un segnale concreto a 5 milioni di poveri, una platea che - ahimè - è raddoppiata rispetto a dieci anni fa, il superamento della legge Fornero, che potrebbe consentire a centinaia di migliaia di persone di recuperare un po' di tempo e di dedicarlo alla famiglia o anche di dedicarlo a loro stessi, e abbiamo messo il fondo per i risparmiatori truffati dalle banche, che abbiamo finanziato con un miliardo e mezzo, una cifra che è 15 volte superiore rispetto allo stanziamento del precedente Insomma, stiamo scommettendo sulle persone. E' qui che nasce il concetto di pace fiscale. È vero, c'è una guerra che tanti poveri cristi stanno combattendo tutti i giorni. Per questo si deve chiamare pace fiscale, perché questa è un'altra possibilità che si dà alle persone che sono inciampate. Non c'è un condono, l'ho cercato bene; non c'è un condono. I condoni li avevamo conosciuti, varati da altri Governi, come nel 2001, quando con lo scudo fiscale si pagava solo il 2,5 per cento sull'importo dichiarato per regolarizzare i capitali, con tanto

di far riemergere i capitali dall'estero. Bene, con questo decreto-legge non c'è spazio per sconti a evasori e furbetti vari. È una pace fiscale, perché - ripeto - ci sono state tante guerre combattute da poveri cristi. Allora noi a questi poveri cristi diamo la possibilità di ripartire, anche per esempio con la cancellazione delle cartelle esattoriali sotto i 1.000 euro risalenti al periodo tra il 2000 e il 2010; così diamo respiro ai piccoli contribuenti e soprattutto evitiamo di perdere del tempo per andare a riscuotere dei crediti vecchi, quel tempo alla vera lotta all'evasione fiscale. Quello sì che è un grande impegno che questo Governo deve assolutamente centrare. Poi abbiamo la rottamazione-*ter*, che estende da due a cinque gli anni entro i quali i contribuenti possono regolare la loro posizione. delle liti pendenti, con cui si va incontro ai contribuenti che hanno ottenuto una vittoria nei confronti dell'Agenzia delle entrate in primo o in secondo grado, permettendo un alleggerimento dei carichi sulle commissioni tributarie; anche qui diamo quindi la possibilità di dedicare tempo alla lotta ai grandi evasori. Con la definizione agevolata del processo verbale di constatazione degli accertamenti, abbiamo dedicato un pensiero e un incontro materiale ai contribuenti, che potranno quindi vedersi scontati sanzioni e interessi, fermo restando il pagamento dell'imposta. Ci dicevate che abbiamo cancellato il *bonus* bebè e invece non è vero che è stato cancellato. Anzi, correggendo alcuni piccoli errori, abbiamo la possibilità

un tema che ci sta talmente a cuore che abbiamo istituito un tavolo dedicato alla lotta al caporalato, per combattere i fenomeni ancora troppo diffusi di sfruttamento dei lavoratori. inoltre prorogato di dodici mesi la mobilità in deroga per i lavoratori delle aziende nelle aree di crisi industriali complesse. Importante è anche il provvedimento che riguarda la sanità e la politica, dire basta alla compatibilità tra il ruolo di Presidente di Regione e quello di commissario straordinario; queste due figure non possono essere sovrapponibili, ma devono essere incompatibili. L'edilizia agevolata è un tema su cui, per fortuna, c'è stato un voto ampio, perché dobbiamo metterci in testa che le periferie sono centrali, non sono un pezzo di città

a chi ha casa in periferia, abbiamo dimostrato di essere loro assolutamente vicini e gli abbiamo dato la possibilità di ripartire. La rete unica delle telecomunicazioni è la grande scommessa infrastrutturale di cui si parla tanto. La digitalizzazione è un percorso, un pezzo di strada che assolutamente dovremo fare, ma che possiamo fare soltanto se scommettiamo realmente sulle tecnologie e sulle infrastrutture tecnologiche. E allora abbiamo gettato le basi per la realizzazione di una rete unica delle telecomunicazioni. Abbiamo scommesso sul futuro; non ci siamo inventati digitali terrestri. Scommettiamo realmente su un qualcosa che farà viaggiare la nostra economia. Per concludere, diamo la possibilità di riordinare proprio questo settore e apriamo la strada alla costituzione di una società unica della rete, alla quale conferire le attuali reti di Tim-Open Fiber. con questo pezzo di strada, che si inserisce in un quadro organico del Governo, abbiamo dato un segno concreto verso quegli operatori economici, verso quelle famiglie che avevano bisogno di attenzione e avevano Questo si inserisce in un disegno più ampio, che sono le proposte di questo Governo. Per tali ragioni su questo decreto-legge il MoVimento 5 Stelle convintamente dice sì.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo ricordare a distanza di qualche settimana dalla loro morte, Stefania Signore e i figlioletti Cristian e Nicolò Frijia di sette e due anni, le tre vittime dell'alluvione che lo scorso 4 ottobre ha colpito tutta la Calabria e in particolare le aree di Crotone, Reggio Calabria e Lamezia Terme. La loro auto è stata travolta da un fiume di acqua, fango e detriti causata dalla troppa pioggia caduta. La macchina di Stefania è stata trovata vuota. La furia dell'acqua ha trascinando i tre passeggeri per 900 metri depositandoli, alla fine, in un fosso di scolo a valle a distanza di 50 metri l'uno dall'altro. Proprio in queste ore si sta consumando un altro tragico evento proprio nella mia città Corigliano-Rossano. Stanotte, infatti, le contrade di Thurio e Ministalla sono state completamente coperte dall'acqua, case comprese, a causa di una nuova esondazione del Crati. L'acqua non riesce a defluire perché i fossi di scolo sono pieni e le zone di rispetto usate per coltivare agrumeti. Solo grazie al lavoro dei Vigili del fuoco e della Protezione civile sono state messe in sicurezza una cinquantina di famiglie. I danni sono ingenti e sono morti anche più di 300 capi di bestiame. Questi casi mettono a nudo come alcuni territori siano martoriati dall'abusivismo edilizio, dalla mancata pulizia dei canali, dalla tombatura dei torrenti. Quando l'acqua aumenta di portata non riesce a defluire e, a causa della piena, fiumi, torrenti e canali straripano, provocando danni e disgrazie. In Calabria non bisogna attendere una nuova tragedia. È necessario che i corsi dei fiumi vengano puliti, che si accertino gli abusi edilizi e si provveda al ripristino dello stato dei luoghi, soprattutto nelle zone a rischio idrogeologico. Noi cittadini di Corigliano Rossano abbiamo ancora negli occhi il tragico evento alluvionale del 2015, quando persone e auto vennero trascinate dalla forza delle acque straripate. Questa estate ci aveva pensato la procura della Repubblica di Castrovillari, con i fermi e i sequestri avvenuti nell'ambito dell'operazione «Flumen Luto», a far vedere come le cose non fossero gestite secondo la legge. Da quest'Assemblea invito ancora una volta il presidente della mia Regione, Oliverio, a sollecitare il soggetto attuatore del rischio idrogeologico affinché si possano intraprendere tutte le iniziative possibili. Gli rinnovo l'invito, già fattogli in occasione dell'allerta meteo lanciata della Protezione civile della Calabria martedì 23 ottobre, quando, con una nota stampa, avevo invitato sia il presidente della Regione Calabria Oliverio, ma anche tutti i soggetti responsabili, come Province, consorzi di bonifica e soggetti attuatori, del rischio idrogeologico ad assumersi le proprie responsabilità e a mettere in atto una serie di misure per gestire i problemi creati dalle esondazioni dei fiumi. Sono diversi i *tornado* che stanno colpendo in questi giorni la Calabria; l'ultimo domenica si è abbattuto sul crotonese, dimostrando come siano in atto importanti variazioni climatiche alle quali bisogna necessariamente far fronte. Bisogna premunirsi e fare prevenzione affinché, *in primis*, fiumi, torrenti e canali vengano puliti e sia attivata la sorveglianza idraulica dei bacini. Solo così non piangeremo altre morti bianche.

e un problema gravissimo, indegno di una Nazione civile come l'Italia. Centinaia di cittadini, che ora sono diventati migliaia, perché con i nuovi mezzi tecnologici è possibile per tutti filmare tranquillamente quello che accade, hanno potuto testimoniare

scene apocalittiche. Sembra di essere in Indonesia o in Cina, nel Fiume Giallo, dove una industrializzazione selvaggia, senza precedenti, ha

venerdì 24 novembre a Ceccano, in provincia di Frosinone, a pochi chilometri da qui. Non parliamo dell'altro emisfero, ma della Valle del Sacco, tra la provincia di Frosinone e la provincia di Roma. Un fiume, il fiume Sacco, noto proprio perché fa parte del SIN (Sito di interesse nazionale),

Sono qui a rappresentare questo incredibile e increscioso episodio, l'ultimo di una serie che sta mettendo a dura prova le nostre popolazioni. La Valle del Sacco è già molto nota proprio perché già inserita nel SIN

ritrovato a seguito della esondazione di centinaia di fusti interrati nel fondo del fiume. Dagli studi risulta che sia entrato nella catena alimentare e, purtroppo, abbia contagiato anche il sangue degli abitanti della zona. Esistono - e sono comprovate - connessione importanti tra l'inquinamento ambientale della Valle del Sacco e la presenza di numerose patologie tumorali.

onorevoli senatrici e senatori, lunedì durante una nota trasmissione televisiva di inchiesta sono emersi alcuni limiti nell'utilizzo dei dispositivi medici che riguardano la registrazione, la tracciabilità e il controllo. Tali

Il professor Romeo, di fronte a delle domande formulate in maniera educata da un giornalista durante un congresso all'estero, dichiarava di aver fotografato lo stesso e, quindi, di aver richiesto informazioni sul suo conto, su suggerimento (farfugliando cose poco chiare) dei parenti, della DIGOS (ricordo che la DIGOS è la divisione investigazioni generali e operazioni speciali della Polizia di Stato), con un atteggiamento minatorio e, a dir poco, inquietante e sicuramente poco consono a un medico, a un chirurgo, a un professore universitario. Il professore avrebbe ottenuto informazioni in ventiquattro ore, meglio di qualunque servizio segreto. Non solo; lo stesso cardiologo affermava di conoscere il direttore di Rai 3, il vicedirettore e i caporedattori di una televisione di Stato. Erano tutti gli amici suoi e persone serie, a suo dire, lasciando intendere al giornalista i rischi a cui si stava esponendo continuando il servizio. Le conoscenze nella Rai si sono dimostrate false, come detto e confermato dai conduttori. A questo punto, davvero spero che anche il resto sia stato solamente millantato. In ogni caso, è inquietante. vero, invece, che il soggetto in questione ha impiantato valvole cardiache senza seguire le linee guida che già dal 2010 impongono agli ospedali di avere un *heart* *team* composto da diversi specialisti che insieme valutano l'appropriatezza. La scienza dice che tali procedure devono essere fatte in determinati pazienti ad alto rischio. Viene, quindi, spontaneo domandarsi a quali soggetti il cardiologo ha impiantato le valvole e come stanno oggi i pazienti. Chi ha deciso gli impianti? Quali sono le complicanze? Dov'era la dirigenza dell'ospedale mentre tutto ciò accadeva, visto non vi era un *heart team* finché i giornalisti hanno chiesto spiegazioni lo scorso ottobre? Lo stesso Romeo ha dichiarato di non aver percepito soldi da una ditta. Falso. Ho chiesto personalmente e ufficialmente mi è stato risposto che dei soldi sono stati dati alla sua unità operativa. Lo stesso Romeo ha dichiarato che la colpa dei prezzi delle valvole è da ricondurre alle ditte che le vendono, che fanno dei prezzi superiori del 300 per cento per il Servizio sanitario nazionale. Falso. Ho chiesto personalmente e i prezzi sono uguali per le strutture private e per il nostro Servizio sanitario nazionale. La verità è una sola: nessuno deve pensare che tali comportamenti possano ritenersi consolidati e impunibili. L'ordine dei medici a cui questo medico è iscritto dovrebbe immediatamente intervenire e lo smesso Ministero dell'interno - immagino avrà da commentare i suggerimenti preziosi della DIGOS, così ben evocati e liberamente esposti. Il Ministro della sanità non potrà esimersi dall'inviare ispettori allo scopo di accertare quanto accaduto. Sarebbe necessaria un'immediata sospensione del cardiologo e di tutta la dirigenza dell'ospedale che non ha vigilato.

di essi nell'ambito di un'università che troppe volte appare sui giornali per condotte poco chiare e censurabili. Queste azioni, non difficili da applicare, rappresenterebbero un punto fondamentale per ridare fiducia ai nostri cittadini nel Servizio sanitario nella ricerca e nell'università. Chi ha sbagliato, questa volta pagherà. Questo è il Governo del cambiamento e una risposta ferma, decisa e inequivocabile verrà data. Lo Stato non è quello descritto dal professor Romeo, quello è

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Comune di Monte San Savino, in Provincia di Arezzo, la notte scorsa, intorno alle ore 4, è stato il teatro dell'ennesimo tragico fatto tragico fatto di cronaca, in cui un onesto cittadino è stato costretto a uccidere per difendere quanto di più sacro esiste: il proprio lavoro e la propria libertà. Fredy Pacini, cinquantasettenne titolare di un'officina ai piedi di Monte San Savino, ha subito stanotte la trentottesima rapina ad opera di due malviventi, tra cui il ventinovenne moldavo colpito poi alla gamba e morto nel tentativo di fuga. Fredy aveva denunciato i continui furti in ogni modo, addirittura gridando la sua esasperazione alle telecamere di Mattino Cinque, che poco tempo fa avevano acceso i riflettori sulla storia di questo cittadino savinese. aveva chiesto di intervenire in modo incisivo per rispondere a una situazione ormai fuori controllo. Fredy chiedeva solo sicurezza per sé e il proprio lavoro. Si è rivolto però a uno Stato che non ha dato le risposte che avrebbe dovuto. Lo Stato, come ha fatto per troppo tempo in passato, ha abbandonato di nuovo un cittadino che chiedeva sicurezza. Fredy dormiva da mesi nella sua officina per difendere la sua unica fonte di sostentamento dalle continue aggressioni di spregiudicati malviventi. Stanotte Fredy è stato costretto a sparare per difendere sé stesso e la sua officina dall'aggressione di due delinquenti entrati con un piccone dalla finestra. Oggi Fredy viene indagato, colpevole di essersi ribellato al trentottesimo rapinatore, da quello stesso Stato cui aveva chiesto protezione. La solidarietà va a Fredy e alla sua famiglia, verso cui lo Stato ha un debito enorme per non aver saputo assicurare la giusta risposta al grido d'aiuto lanciato. decreto sicurezza, nelle prossime settimane la Camera dei deputati sarà impegnata a approvare il nuovo testo in tema di legittima difesa, già approvato in Senato nell'ottobre scorso. Dimostreremo a Fredy, alla sua famiglia, alla comunità savinese esasperata da un intollerabile clima di paura

*(M5S)*. Signor Presidente, non è la prima volta, purtroppo, che intervengo in quest'Aula per parlare di mafie e, in particolare, di quelle operanti in provincia di Foggia. Si tratta di sodalizi criminosi che nel giro di trenta-trentacinque anni circa si sono costituiti in un'unica entità definita dagli inquirenti e dal Procuratore nazionale antimafia la quarta mafia italiana. Questa mafia, purtroppo, è diventata ormai *leader* in alcuni traffici e si distingue per ferocia, sfrontatezza, aggressività e stretti vincoli familiari, il che la rende più impermeabile al lavoro e alle indagini degli inquirenti. Questa quarta mafia ha compiuto più di 300 omicidi negli ultimi anni, l'80 per cento dei quali rimasti impuniti - questo è quello che ci dice il CSM - e purtroppo negli ultimi dieci giorni si sono verificati altri due omicidi: uno a Foggia, una decina di giorni fa, in una stazione di servizio dove ha perso la vita un pregiudicato e uno a San Severo, sabato scorso, quando in pieno centro si è realizzato un inseguimento di un altro pregiudicato che

che comandano loro e ammazzano chiunque, quando e come vogliono loro. È la risposta criminale che queste organizzazioni danno al tentativo dello Stato di contrastarle. Noi crediamo che lo Stato debba innalzare sempre più il livello di contrasto messo in campo sia dal precedente Governo, sia da quello attuale che rispettivamente hanno istituito il reparto prevenzione crimine a San Severo e lo squadrone elitrasportato cacciatori di Puglia che avrà stanza nell'aeroporto militare Questi due ultimi omicidi devono però farci capire che siamo ancora molto lontani dall'aver sconfitto queste mafie. Ora dobbiamo operare il massimo sforzo per togliere linfa vitale a questi criminali, dobbiamo dotare il territorio di ancora più mezzi, più Forze dell'ordine e più polizia giudiziaria, più magistrati. A quest'ultimo proposito, ho presentato qualche settimana fa un disegno di legge per l'istituzione a Foggia della sezione distaccata della Corte d'appello di Bari e soprattutto per l'istituzione della Direzione distrettuale antimafia a Foggia e spero proprio che questa proposta riceva l'attenzione di tutte le forze politiche. Siamo infatti convinti che avere presidi giudiziari specializzati che hanno sede proprio nei luoghi in cui queste mafie spadroneggiano consentirà un migliore contrasto alle attività criminose. *(Applausi